onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione, con modificazioni,

oggi discutiamo un provvedimento che tocca temi cruciali, che affronta lo sviluppo e la protezione ambientale, l'autonomia energetica del nostro Paese e le difficoltà dei cittadini relative al caro bollette e alla crisi energetica. Speravamo che al Senato venisse concesso un tempo adeguato, ma ci troviamo, ancora una volta, a ratificare il lavoro della Camera, visto che è stata posta la questione di fiducia. poiché si poteva evitare il decreto-legge con un accordo preventivo sui tempi di approvazione. Nonostante ciò il decreto-legge ha il merito di dare un forte impulso al tema delle comunità energetiche e supera finalmente il colpevole ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi. Queste comunità stimolano l'uso di energie rinnovabili, promuovendo la sostenibilità ambientale e una prospettiva energetica più resiliente. Inoltre supportano l'indipendenza energetica a livello locale e rafforzano il senso di comunità, mostrando come un approccio collettivo all'energia possa portare benefici sia economici che ambientali. Questo rappresenta un passo importante verso l'autonomia energetica che il Paese deve perseguire. In poco più di un anno l'Italia è riuscita a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, ma un Paese è veramente libero solo se riduce la quota di importazioni del proprio fabbisogno energetico. È essenziale che la politica energetica non rimanga bloccata sul presente, ma consideri anche le fonti e le tecnologie future. Sono in corso di sperimentazione tecnologie che potrebbero trasformare completamente il panorama della produzione e dell'approvvigionamento energetico nei prossimi decenni. Occorre una politica che guardi oltre il 2050, che incentivi e sostenga l'innovazione tecnologica nel settore energetico, coniugando autonomia, sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente. Rimane il rammarico per non aver avviato un serio confronto con l'Europa sulla fine del mercato tutelato. Pratiche commerciali aggressive e scorrette stanno danneggiando i consumatori che subiscono aumenti legati più a pratiche speculative che a reali incrementi delle materie prime. Il mercato dell'energia rischia di diventare una giungla piuttosto che un ambito concorrenziale a beneficio del cittadino consumatore. Per le stesse ragioni noi pensiamo che con l'Europa vada affrontato il tema delle piccole derivazioni idroelettriche, che sono l'altro lato della medaglia delle comunità energetiche o potrebbero esserlo. Esse nascono per essere al servizio del territorio, molte di loro non hanno e non avrebbero neppure mercato; sarebbe quindi giusto che esse continuassero a svolgere la loro funzione fuori dall'ambito del mercato e fuori dall'obbligo delle procedure di gara. Concludendo, Presidente, pur riconoscendo lo sforzo compiuto e non entrando nel merito degli altri temi oggetto del provvedimento, percepiamo comunque la mancanza di una strategia a lungo termine, in particolare per quanto riguarda sia le energie rinnovabili che la situazione attuale vissuta da milioni di italiani con la fine del mercato tutelato. Essendo stata posta la questione di fiducia, il Gruppo per le Autonomie non potrà esprimere un voto completamente favorevole al provvedimento.

la politica energetica è un aspetto fondamentale delle politiche nazionali, perché è l'intersezione di diverse politiche. La politica energetica è essenzialmente politica industriale, è politica ambientale ed è politica che attiene alla sicurezza, nella misura in cui la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è uno degli aspetti fondamentali delle relazioni geopolitiche internazionali e della tutela degli interessi nazionali, come purtroppo ci dimostra drammaticamente il caso del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, che è un territorio di passaggio del gas che proviene dalla Russia. Tuttavia questo provvedimento, che oggi è in fase di votazione finale al Senato, non contiene quella visione di politica energetica che un Paese forte e industrialmente importante come l'Italia meriterebbe. Questo provvedimento è una legge contenitore, all'interno della quale si buttano tante cose eterogenee, ma senza una visione di politica energetica. Ci sono diversi aspetti positivi del provvedimento, ma ci sono anche alcune contraddizioni, che noi cerchiamo sempre, come Azione, di valutare e di stigmatizzare per uscire dal furore ideologico ed entrare nel merito del provvedimento. Faccio l'esempio dell'*offshore* eolico galleggiante.

Io inviterei i colleghi e il Governo a dirci quanti *offshore* eolici galleggianti ci sono in Europa in questo momento: pochissimi. E perché? Perché è difficile pensare che questa tecnologia possa essere davvero competitiva nel mar Mediterraneo, dove c'è molto vento e dove le acque sono in genere più profonde. è solo un piccolo esempio di alcune cose che probabilmente, se fossero state oggetto di interlocuzione tra maggioranza e opposizione, avrebbero portato a un miglioramento del testo del provvedimento e che oggi invece, con la posizione del voto di fiducia, avete deciso di blindare. Penso al tema del nucleare. Sento che la maggioranza sostiene con orgoglio di aver fatto uscire il tema del nucleare da un tabù italiano. Vi ricordo che ieri, nella prima discussione all'Assemblea nazionale francese, il nuovo *premier* Attal ha parlato invece di orgoglio francese nella produzione di nucleare. Qui in Italia stiamo cercando di uscire da un tabù ideologico, laddove i nostri cugini d'Oltralpe dichiarano con orgoglio che è grazie al nucleare francese se le aziende e le imprese in Francia pagano competitivamente molto di meno rispetto alle imprese italiane e ad altre imprese europee. Anche qui c'è una contraddizione, qui c'è una contraddizione, quella di non riconoscere che moltissime delle forze politiche presenti in questo Parlamento hanno votato, all'interno del Parlamento europeo, una normativa sulla tassonomia *green* che riconosce il nucleare di ultima generazione come una fonte *green*. *green*. Lo dico rispetto a chi oggi ha pudore sul tema dell'energia nucleare di ultima generazione, laddove invece dovremmo aiutare questo Paese; noi cerchiamo di farlo, con tante iniziative per cercare di raccogliere le paure che gli italiani hanno su alcuni argomenti, come il tema delle scorie e quello della destinazione degli impianti. Abbiamo visto che il Governo ha aperto al tema della autocandidatura degli impianti. Io credo, però, che se noi non riusciamo, non a parlare di questo tema con pudore, ma a parlarne con coraggio e con forza, rischiamo di non dare concretezza a quei timidi

Vorrei sottolineare che alla Camera era stato presentato da Azione un emendamento afferente a Terna ed afferente al conflitto di interessi tra chi gestisce la rete e chi definisce la strategia energetica. Noi crediamo che su questo tema sia importante, proprio sulla base del principio della separazione tra chi pianifica la rete e chi la gestisce, avere una posizione chiara, strategica e priva di conflitti di interessi.

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, era molta aspettativa per questo decreto, che avete tenuto nel cassetto per molto tempo. In particolare, gli operatori e i cittadini aspettavano ben due provvedimenti:

sulla politica energetica.

è attraccata la prima nave. Infatti con una emergenza energetica come quella che ha vissuto il nostro Paese e con la guerra tra Russia e Ucraina che ancora non vede una fine e quindi con la privazione del gas russo, in attesa che le rinnovabili

si semplificano le norme per avere i rigassificatori, poi bisogna aumentare le tasse per le energie rinnovabili. Bisogna avere una politica d'insieme, che preveda

trovare il nostro gas. Sempre a parole, sembrava che fosse questione di giorni, dopo che il Governo Meloni era entrato in carica, perché finalmente la politica dei no venisse sconfitta. no venisse sconfitta. Invece non c'è un'azione che riguardi il nostro gas. Nel frattempo, per fortuna, tra il Governo Draghi e il Governo Meloni, quello che viene chiamato il Piano Mattei, che riguarda la parte energetica, è stato realizzato da una nostra società, l'ENI, che ha fatto accordi con i Paesi nordafricani per avere il gas e sostituire quello russo, ma tutto questo non ha una base omogenea.

*partner* di ricerche europee e internazionali sul nucleare di nuova generazione, nucleare che inquina di meno e provoca meno scorie.

raccoglie la sollecitazione del Capogruppo, seppure data un po' bruscamente. Prego,

quella della Camera, e non un approfondimento al Senato. Ieri non siamo riusciti neanche a dare il mandato al relatore. Abbiamo analizzato molto velocemente, con pareri che non erano neanche pienamente a conoscenza del Governo, più o meno 12 ordini del giorno. Secondo me questo Paese merita un po' di più, merita una strategia vera sull'energia che ad oggi, non emerge dalle parole e dagli atti del ministro Pichetto Fratin, non emerge dalle politiche del ministro Urso e non emerge dalle politiche del Governo Meloni. Non emerge da questo decreto-legge, che è l'ennesimo decreto sull'energia; fosse il primo si direbbe che è un esercizio di stile, ma non è un esercizio di stile, perché è l'ennesimo decreto-legge senza avere una strategia di insieme e di visione. In particolare, cito due delle materie che i cittadini e gli operatori speravano di trovare in questo decreto-legge e non ci sono, a dimostrazione di quello che stavo dicendo. Per quanto riguarda il libero mercato, noi siamo favorevoli e sappiamo che una libera concorrenza servirà anche in futuro a ridurre i prezzi, ma bisognava fare dei passi prima di arrivare al libero mercato per i cittadini, che non sono stati compiuti. In particolare, una vera analisi dei venditori: c'è un elenco di 638 soggetti che sono autorizzati a fare offerte ai cittadini. Ma secondo voi ci sono 638 operatori che si occupano di energia in questo Paese? A me non sembra. Vuol dire che ci sono dei prestanome e che sicuramente le truffe sono dietro l'angolo:

a chi dice loro «ti faccio risparmiare, vieni con noi». Noi avevamo bisogno di tutelare non solo le persone fragili, che continuano a essere nel mercato tutelato, ma anche le persone che tecnicamente, per un motivo di età, fragili non sono, ma hanno il diritto di avere operatori veri e non degli operatori truffa. In secondo luogo, l'idroelettrico: ne ha già bene parlato ieri il collega, capogruppo Enrico Borghi. La tolgo dall'imbarazzo:

iniziava il periodo della siccità, anche se era inverno, dare a libera gara le concessioni idroelettriche e in un solo colpo dare a libera gara acqua ed energia era un controsenso. All'epoca Fratelli d'Italia era con noi,

che se ci avessimo ripensato, come hanno fatto la Francia, il Portogallo, la Spagna, la Germania, la Norvegia, cioè tutti i Paesi europei,

non dice assolutamente questo, ma innanzitutto dice che i grandi impianti idroelettrici sono reti sensibili e come tali vengono gestiti dal Paese. È per quello che quando c'era il Governo Draghi noi chiedemmo che quella materia fosse trattata come *golden power*, che fosse emanato

c'era una progressiva messa a gara con un accordo Stato-Regioni e invece qui ognuno è battitore libero e fa un po' quel che gli pare: ci sono Regioni che hanno messo a gara da due anni i loro impianti e non hanno avuto frutto e ci sono ricorsi al Consiglio di Stato e al Tar, perché è una materia troppo sensibile. Soprattutto, non riesco a capire perché, invece di rendere appetibile a società straniere di energia - molti mi dicono che Edison esiste già in alcuni impianti ed è verissimo - rischiamo di regalare quegli impianti ai fondi di speculazione. Voglio vedere, quando ci sarà la prossima siccità e dovranno immettere l'acqua nei fiumi,

altro che sovranità italiana: noi rischiamo di svendere il nostro patrimonio energetico e il nostro patrimonio di acqua. Per questi motivi, voteremo con profonda convinzione contro la fiducia a questo Governo.

Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, non nascondo una certa insofferenza nel dover dichiarare di nuovo la contrarietà del mio Gruppo anche a questo provvedimento sull'energia che, oltre ad essere antistorico e anacronistico, risulta sprezzante delle conquiste che sono state raggiunte con grande fatica in tema climatico, sia a livello europeo che internazionale, tanto più che proprio il mese scorso ho avuto il privilegio di assistere personalmente ai lavori della COP28, conclusasi con la firma di uno storico accordo che ha evidenziato per la prima volta nero su bianco l'improrogabile necessità di fuoriuscire dall'utilizzo dei combustibili fossili entro il 2030 e al contempo il bisogno di triplicare la capacità di produzione di energia rinnovabile, un impegno internazionale firmato incredibilmente da 196 Paesi, tutti concordi sull'urgenza di garantire con tutti gli sforzi possibili un futuro al nostro pianeta, oggigiorno devastato ad ogni latitudine dai tragici effetti della crisi climatica, alimentata anche dall'utilizzo delle fonti fossili, accordo firmato anche dall'Italia. Il tempo per decidere se sia opportuno o no perseguire l'obiettivo di transizione energetica è scaduto. Non si può più discutere sul se, ma sul quando e come attuarla, così da garantire per noi stessi e per le future generazioni la possibilità di vivere in un ambiente sano, senza la costante minaccia di perdere anche la propria vita. Lo sanno bene le piccole isole del Pacifico, come Samoa, che potrebbero scomparire a breve per l'innalzamento repentino del livello dei mari. Una condizione drammatica globale che sta flagellando anche l'Italia e la sua economia e che non possiamo più ignorare. Pertanto, proprio dinanzi all'urgenza di un cambio di passo siglato anche dall'accordo di Dubai, alla coesione di Paesi geograficamente, culturalmente e politicamente così lontani (ricordando che anche i Paesi arabi, storici produttori ed esportatori di combustibili fossili, stanno investendo enormi capitali in energie rinnovabili), l'Italia, con il suo attuale Governo, invece di approfittarne, retrocede, si disallinea, si deresponsabilizza e si nasconde, a questo punto direi vigliaccamente, firmando accordi internazionali ad alto livello, per poi tornare in Italia e continuare a varare politiche dannose e anacronistiche, che continuano ad andare a braccetto con il fossile e sbarrano la porta al progresso, al presente, già travagliato dal susseguirsi di eventi climatici estremi, e al futuro. È desolante vedere il proprio Paese arretrare rispetto all'opportunità di affrontare in modo sinergico e strutturato una problematica seria e urgente come quella del cambiamento climatico, condizione che tocca da vicino la vita, la salute e il benessere economico dei cittadini. Eppure questo Governo dovrebbe saperlo bene, visto che anche nel provvedimento in esame prevede degli aiuti, che io chiamerei "toppa", per le comunità emiliane e toscane che, dopo i disastrosi eventi meteorologici verificatisi da maggio 2023 in poi,

fotografa perfettamente il momento parossistico che sta vivendo il Governo Meloni, così confuso e diviso tra la sua apparente veste diplomatica, che sfoggia con ipocrisia in tutti gli appuntamenti internazionali (la COP, il G7 e il G20) e la sua reale vocazione politica retrograda, dannosa e colonialista, votata all'esasperato sfruttamento e approvvigionamento di combustibili fossili sia all'estero che a casa propria. stesso dualismo politicamente ingannevole che ripropone in questo testo, dove sapientemente nasconde, tra qualche magra disposizione apparentemente orientata alla sostenibilità, la volontà di rilanciare l'attività di estrazione degli idrocarburi non solo nei siti già attivi, ma anche in ambienti marini questo modo, fingendo di sostenere la produzione da fonti di energia rinnovabile, in realtà aumenta in modo preoccupante gli incentivi economici per i settori gasivori, ossia per quei comparti industriali altamente dipendenti dal consumo di gas. Aprire al rilascio di concessioni per coloro che intendono costruire nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, oltre ad essere moralmente deplorevole, ci autodelegittima come Paese, rendendoci incoerenti e sprezzanti, non solo dinanzi agli impegni internazionali ed europei, ma anche al cospetto della nostra Costituzione, che all'articolo 9 tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi naturali che lasceremo in eredità alle future generazioni. Ci chiediamo come sia possibile che questo Governo, piuttosto che approfittare delle enormi opportunità di sviluppo economico e occupazionale offerte dalle fonti rinnovabili, preferisca ancora una volta agevolare quei settori altamente inquinanti che, oltre a danneggiare la salute dei cittadini e dell'ambiente, sono senza futuro nella prospettiva Si utilizzano soldi pubblici per costruire impianti obsoleti di incenerimento in Sicilia, di conservazione e gestione dei rifiuti radioattivi; strutture che da circa vent'anni vengono considerate dalla Comunità europea e internazionale come residuali nella piramide del ciclo dei rifiuti. scelte inquinanti e irrispettose della tutela ambientale. Insomma, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, lo stesso mare del nostro stupendo e invidiato Paese che non risparmiate di trivellare. Nella giornata parlamentare della COP28, organizzata dall'Unione interparlamentare e dal Consiglio nazionale federale degli Emirati Arabi Uniti, a cui hanno partecipato parlamentari provenienti da settantasei si è sottolineato il ruolo cruciale che svolgono i parlamentari nell'esercizio di indirizzo nei confronti dei nostri Governi. È per tale ragione che in quest'Aula, anche in questa occasione, mi rivolgo alla maggioranza e al Governo - anche a lei, signor Sottosegretario - ribadendo l'importanza di agire e dare fondamento agli impegni presi, vincolandoli a politiche coerenti che sappiano concretamente garantire una transizione ecologica, giusta, equa e sostenibile. Pretendere di continuare a vivere in modalità *business as usual* non è più un'opzione. È arrivato il momento che ne prendiate coscienza. Il nostro futuro dipende dal nostro presente

il decreto-legge in esame è un provvedimento strategico sul tema dell'energia in Italia, fondamentale per la decarbonizzazione, l'economicità e la sicurezza nella produzione dell'energia. provvedimento che si è ulteriormente arricchito durante l'*iter* parlamentare alla Camera con un approfondito esame che è stato seguito puntualmente dal ministro Gilberto Pichetto Sono stati approvati cento emendamenti che hanno aggiunto sedici articoli e decine di commi, con il contributo di Forza Italia, della maggioranza, ma anche dei deputati di minoranza. Peraltro, l'esame di merito ha seguito un vasto ciclo di audizioni degli *stakeholder*, sia pubblici che privati, che hanno dato il proprio sostanziale contributo assieme a diversi esperti del settore. Possiamo quindi affermare che il provvedimento ha avuto un esame approfondito e senza alcuna preclusione ideologica. le opposizioni sostengono che questo sia un decreto-legge vuoto, senza nessuna novità su transizione ecologica, fonti rinnovabili, ambiente, decarbonizzazione. Allora vediamo insieme cosa contiene questo decreto vuoto. Due sono gli obiettivi principali: promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili e sostenere le imprese a forte consumo di energia. previste altre misure, ad esempio a sostegno dell'edilizia; disposizioni per la ricostruzione dei territori alluvionati del 2023 e in favore dei territori umbri colpiti dal sisma; disposizioni per l'accesso al fondo di solidarietà per le imprese agricole, per il riutilizzo dei materiali di drenaggio, per gli impianti di illuminazione pubblica. Inoltre voglio ricordare che, grazie a Forza Italia, sono state introdotte norme nell'ambito del libero mercato dell'energia: siamo cioè intervenuti per assicurare il minor impatto e le maggiori garanzie possibili ai clienti finali, sia famiglie che imprese. L'approvazione del cosiddetto *electricity release* serve a garantire un sostegno per gli energivori elettrici, promuovendo al contempo lo sviluppo di nuovi impianti da fonti rinnovabili. presente anche una misura a sostegno delle imprese cosiddette gasivore, che potranno acquistare il gas a un prezzo vantaggioso rispetto alle quotazioni di mercato. Vengono dichiarati interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti tutte le opere finalizzate alla costruzione di rigassificatori. È stata raddoppiata la dotazione del Fondo per la transizione energetica del settore industriale, proprio per sostenere la competitività delle nostre imprese nei settori maggiormente esposti al rischio di rilocalizzazione. Sono state prorogate al 31 dicembre 2026 le concessioni geotermiche, consentendo di rimodulare, a determinate condizioni, l'esercizio delle concessioni per un periodo fino a vent'anni.

Sono state introdotte anche molte semplificazioni: semplificazioni alle autorizzazioni per realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, eoliche e solari; semplificazione della procedura di smaltimento dei pannelli solari esauriti; semplificazione all'accesso agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area colpita dagli eventi sismici del 2016. previsto un innalzamento delle soglie per la sottoposizione dei progetti a valutazione ambientale, semplificando le procedure autorizzative per le opere di connessione alla rete elettrica per gli impianti da fonti rinnovabili. Vengono definiti più puntualmente gli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole; così come viene agevolata la produzione di energia elettrica e calore da biomasse, solide e gassose. Inoltre, sono state introdotte disposizioni in materia di installazione di impianti a fonte rinnovabile in siti oggetto di bonifica. È stato istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto a tener conto della peculiarità della filiera. cito le norme per la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio e in corso di realizzazione, tema sul quale Forza Italia era già intervenuta in Senato recentemente con una serie di agevolazioni. È stata prevista la procedura per l'individuazione di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione, alla produzione e all'assemblaggio di piattaforme eoliche galleggianti *offshore*. Le agevolazioni in materia di accisa, previste per il gasolio, si applicheranno anche al biodiesel, con lo scopo di incentivarne l'utilizzo. Vi sono norme anche in materia di stoccaggio geologico di CO2, il cosiddetto *carbon capture and storage*, che puntano a centrare gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030. Viene rifinanziato per il 2024 anche il Fondo italiano per il clima, per sostenere gli interventi a favore di soggetti privati e pubblici. altro che decreto-legge vuoto! Un corposo insieme di norme che persegue gli obiettivi europei che l'Italia ha fatto propri, per un Paese avviato verso la decarbonizzazione e un sempre più spiccato indirizzo nazionale alla produzione di energia pulita e rinnovabile.

Vedete: sono tutti risultati positivi, che aumenteranno con gli effetti benefici di questo decreto-legge. Come potete rilevare, la tutela dell'ambiente, la decarbonizzazione, l'impiego di fonti rinnovabili non sono temi in esclusiva alle sinistre, anzi. C'è chi si riempie la bocca con questi obiettivi e poi ci siamo noi di centrodestra che li realizziamo. Per questo il Gruppo Forza Italia

poter almeno discutere i nostri emendamenti - quindi è l'ennesimo atto di prepotenza da parte di questo Governo - in realtà, sotto un falso nome - perché di sicurezza energetica e fonti rinnovabili c'è pochissimo o nulla - è un provvedimento sulle energie fossili inquinanti e costose. Infatti prevede nuove trivelle, con il rischio subsidenza, che andranno a mettere in serio rischio le nostre coste.

coloro che vendono le energie, causando nuovi extraprofitti, che tanto piacciono a questo Governo. Il provvedimento prevede poi lo stoccaggio di rifiuti nucleari in aree non idonee. Voi, che volete fare una ventina di centrali nucleari, non riuscite a trovare un piccolo deposito di scorie nucleari in tutto il Paese avete addirittura aperto alle aree non idonee la possibilità di autocandidarsi. *(Applausi)*. Ma vi rendete conto? Siete alla frutta.

un Governo che non vuole la transizione energetica e che sta favorendo chiaramente le *lobby* dell'energia. Penso che questi decreti non li scriviate manco voi, ma vengano scritti direttamente dalle *lobby* dell'energia.

Avete anche sancito il nuovo Piano Mattei. Ma cosa andate a fare in Africa? Con tutti i danni che state facendo in Italia, volete andare anche in Africa a farne altri?

Facciamo le piante che produrranno olio e poi prenderemo una nave cargo, alimentata da fonti fossili, per portarlo alla bioraffineria di Gela, che consumerà energia fossile, per produrre biocarburanti. Vale la pena utilizzare direttamente i combustibili fossili, perché per produrre un litro di biocarburante a volte ne servono due di fonti fossili. È quindi un'operazione di *greenwashing* che serve solo per fare speculazione economica nei Paesi poveri. I biocarburanti non servono a nulla, non è energia pulita. Il Piano Mattei quindi è un piano di aria fritta. Io credo che anche Mattei si stia rivoltando nella tomba, perché lui guardava al futuro e oggi il primo che avrebbe capito che le fonti rinnovabili sono il futuro sarebbe stato proprio Enrico Mattei. Avete anche abusato del suo nome: era una persona lungimirante e sicuramente oggi, se fosse vivo, saprebbe benissimo che le fonti fossili sono arrivate al capolinea. Non considerate quindi i costi economici; se avete cinque miliardi e mezzo da spendere, perché non facciamo un grande piano per solarizzare tutti gli edifici del nostro Paese, tutti i capannoni industriali e i parcheggi?

Governo condividesse di più, perché anche loro non sanno cosa volete fare in Africa. gli esponenti dei Governi africani, probabilmente la Meloni abbia riferito cosa vuole fare in Africa ai comici russi. *(Applausi)*. È molto probabile che sia successo questo, perché anche gli africani non sanno cosa volete andare a fare in Africa. Evidentemente voi volete far sopravvivere le fonti fossili, le *lobby* delle fonti fossili, ma non state facendo l'interesse del nostro Paese. Voi qui non dovete fare l'interesse delle aziende che producono, vivono sull'energia fossile e hanno interesse a mantenere questo sistema perché fanno dei profitti. Voi dovete fare l'interesse del nostro Paese che è uno solo: produrci da soli

a parità di costo, l'energia rinnovabile e l'energia solare costano due, tre centesimi a kilowatt, anche dovendo fare dei sistemi di accumulo, potremmo al massimo arrivare a 6-7 kilowatt rispetto ai 30-40 kilowatt dell'energia fossile, includendo lo stoccaggio di CO2, l'esternalità e i costi di produzione. Non parliamo dell'energia nucleare, perché non avete nemmeno un sito per fare i depositi di scorie. Oggi i dati scientifici ci dicono che l'energia nucleare, senza il costo del trattamento delle scorie, si attesta sui 16 centesimi a kilowatt. Questi sono i dati. Allora qual è la verità? La verità è che questa energia pulita non piace a chi oggi vende l'energia e vuole mantenere dei profitti sulla sua vendita ai cittadini, perché autoprodursi l'energia è conveniente per i cittadini, ma non per le *lobby*. *(Applausi)*. Questa è la verità!

È evidente che non ha senso, come detto, per motivi di bilancio energetici produrre biocarburanti in Africa. Non ha senso nemmeno dal punto di vista occupazionale, perché l'Africa è enorme, servirebbero milioni di posti di lavoro; non sarà qualche ettaro di colture energetiche a risolvere il problema dei flussi.

la ringrazio per la sensibilità di aver rispettato un pochino la fatica di arrivare qua. Devo dire che, quando ho sentito giustamente denunciare la nostra amica in carcere con i ceppi, io dico, senza fare vittimismo, che esistono ceppi che alcuni Paesi mettono alle persone in corso di indagine ed esistono Paesi civili come l'Italia, per la quale ho combattuto molto, che mettono ceppi invisibili o visibili come quelli delle barriere architettoniche, di traffico e di movimento. Persino in questa Aula, per me sacra, qualche volta mi sento un po' in difficoltà, perché non trovo la posizione giusta per stare correttamente io e non disturbare gli altri. Quindi, ho colto con molto favore la sua sensibilità di darmi il tempo di riadattarmi all'Aula. Continuo - grazie a lei, Presidente, colleghi e colleghe - a dire che l'energia

rivolti al gruppo e hanno cominciato a identificarsi come famiglia solidale proprio intorno al fuoco, intorno al calore, intorno alla difesa dagli animali orribili di quel periodo. Da quel momento l'energia non è stata solo l'agente e il motore del nostro sviluppo, ma è stata anche un momento di rappresentazione delle nostre civiltà. Certo, in questi decenni non abbiamo rispettato la logica, non abbiamo rispettato l'ecosistema e adesso ne paghiamo le

se non per difendere le idee o le persone che vanno difese, e va dato anche spazio di critica e di cittadinanza. Qualche volta, però, mi va di fare polemica, polemica terapeutica spero. Negli interventi di ieri e di oggi delle opposizioni io colgo, con tutto il rispetto - sono stato una vita all'opposizione e ne so qualcosa qualcosa - un nervosismo e, se vogliamo, un doppiopesismo che non considero degno di questa Aula. riferisco al grande successo del Presidente del Consiglio proprio in questa Aula, l'altro ieri, quando il mondo africano ha sentito finalmente non di vecchio e di neo-colonialismo, ma la volontà di fare insieme, la volontà di condividere una scelta comune di crescita per una crescita comune,

Giorgia Meloni ha realizzato con il suo Governo, con il Piano Mattei e con l'Africa, le premesse per superare vecchi e nuovi colonialismi e vecchie e nuove forme di sfruttamento. Questo credo che irriti qualcuno di voi e ciò mi dispiace, perché il percorso condiviso, tra chi dà e chi riceve, ma facendo le cose insieme, è l'unico modello di sviluppo. Dice ciò chi, per poco tempo, è stato, oltre che Ministro della famiglia, anche delegato all'immigrazione. E già allora introdussi misure che ancora ci fanno essere orgogliosi: il diritto alla cura, il diritto all'istruzione dei minori. Io credo che in questo clima, di rifiuto delle realtà, anche il provvedimento del quale parlo questa mattina abbia un senso solo se

perché non mi piace dare la colpa a chi c'era prima, ma certamente comportamenti irresponsabili per decenni hanno prodotto quello che c'è adesso. adesso. Questo provvedimento non è la lista della spesa dei sogni e dei miracoli. È un provvedimento complicato, che prevede una tempistica che forse a qualcuno può sembrare eccessiva, che prevede il rispetto delle aziende e dei cittadini. Non contiene la soluzione immediata per tutto, non è il sogno che diventa realtà. C'è un percorso serio, scientifico, politicamente accettabile da tutti, anche fuori dall'Italia, per uscire dal carbone, per uscire dalle energie avviene ma senza creare povertà, perché poi la pagheremmo in altri modi; senza creare regressi industriali, senza creare disagio nelle nostre famiglie,

di ogni giorno nella difficile normalità, danno esempi di pazienza, di coraggio, di creatività.

certamente pulita, ma efficiente. Lei sa, signor Presidente, che esistono decine di migliaia, milioni di persone che, attraverso l'energia, possono mantenersi in vita? Purtroppo, finché la scienza si preoccuperà più di costruire cannoni sempre più perfetti e non strumenti di terapia e cura per persone con disabilità grave e ingravescente, queste persone, senza l'energia, continueranno

ai colleghi e alle colleghe, ai membri del Governo, così pazienti rispetto a certe intemperanze, e a lei, signor Presidente, così gentile nei miei confronti, che io voterò in maniera serena questo provvedimento, cercando di dimostrare, anche con le parole, al di fuori dell'Aula, che non si può avere tutto e subito. Non si possono promettere miracoli

rappresentanti del Governo, dopo il sì della Camera dei deputati oggi siamo chiamati ad approvare in via definitiva un provvedimento che definirei strategico per il nostro Paese, incentrato sulla promozione della sicurezza energetica dell'Italia, ma in forma *green*, attraverso un potenziamento delle fonti rinnovabili e il sostegno alle imprese energivore e con un occhio anche alle popolazioni colpite dalle alluvioni delle scorso Quanto la nostra dipendenza energetica da altri Stati sia drammatica e possa essere per noi dannosa è emerso purtroppo con tutta la sua forza dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. E da allora scontiamo la nostra dipendenza con un'impennata dei prezzi dell'energia e del gas che incide pesantemente sulle famiglie, ma anche sulle nostre imprese. Da allora abbiamo iniziato a lavorare, sin da subito in maniera anche intensa, come maggioranza e come Governo su più fronti, partendo innanzitutto dai sostegni ai cittadini per difendersi dal caro-bollette e mitigare i costi

intervenuti anche con misure dirette agli enti e alle imprese, come la possibilità per i Comuni di pianificare le politiche energetiche locali, la premialità per le imprese che coprano il 50 per cento del loro fabbisogno con energia verde, la tassa sugli extraprofitti:

tutti - abbiamo stanziato finora 35 miliardi di euro, che - ne siamo convinti - sono stati fin qui utili e preziosi. Ancora, questo provvedimento si occupa di quei milioni di utenti domestici che si servono ancora del mercato tutelato e che devono passare a quello libero. Per la metà di quelle persone ritenute vulnerabili stabiliamo che possano continuare a usufruire di forniture a prezzi calmierati, mentre per tutte le altre famiglie introduciamo misure che possano garantire loro la massima trasparenza, le necessarie informazioni e le migliori condizioni per passare al mercato libero. Ovviamente questi interventi da soli non bastano e parallelamente, quindi, abbiamo continuato a lavorare su interventi di tipo strutturale, con i quali il Governo mira a rendere autonoma l'Italia dal punto di vista energetico. Ancora una volta ci siamo trovati a dover porre riparo alle macroscopiche mancanze di chi ci ha preceduto e che non solo non ha pensato e attuato politiche che potessero aiutarci a raggiungere l'indipendenza energetica, ma ha, viceversa, perfino potenziato la nostra dipendenza, legandoci a doppio filo ad alcuni Stati e portandoci alla complicata situazione in cui oggi ci troviamo. *(Applausi)*. E hanno anche oggi l'ardire di criticare il lavoro di questo Governo. Mi permetto di dire che forse questo provvedimento Mi permetto di dire che forse questo provvedimento non l'hanno letto attentamente. Noi stiamo intervenendo per far sì che il Paese possa pian piano provvedere autonomamente a coprire il proprio fabbisogno energetico, sia per consentire a tutti di accedere all'energia a prezzi adeguati e che questi prezzi possano stabilizzarsi stabilizzarsi al ribasso, sia per garantire e anzi potenziare la competitività delle nostre stesse imprese a livello internazionale. Per raggiungere questi obiettivi non possiamo non passare per l'implementazione delle fonti di energia rinnovabile, contemperando in tal modo l'esigenza di garantire la sicurezza energetica con quella di rispettare la sostenibilità ambientale, e cioè un bilanciamento di questa esigenza con la transizione *green*. Quindi, prevediamo incentivi per le imprese energivore perché installino impianti fotovoltaici ed eolici, quindi fonti rinnovabili, dando loro un arco di tempo anche abbastanza lungo, fino al 2030, sufficiente per poter programmare i necessari interventi. Nell'attesa che i nuovi impianti diventino operativi, prevediamo anche un meccanismo di sostegno, per cui le imprese potranno chiedere un'anticipazione di parte dell'energia prodotta dagli impianti stessi per continuare l'attività, ma anche in maniera conveniente. Tuttavia, il fotovoltaico e l'eolico non sono e non possono essere da soli sufficienti, come ha sottolineato tra l'altro nei giorni scorsi lo stesso loro vice ministro Gava. Quindi, apriamo ad altri tipi di approvvigionamento, le cui necessità sosteniamo da tempo, anche come e soprattutto come Gruppo Lega. Mi riferisco innanzitutto al nucleare: come ben si sa, per noi il nucleare di ultima generazione è la strada migliore per poter avere energia pulita e sicura a basso costo. Per riprendere questa strada, quindi, diamo la possibilità ai Comuni di autocandidarsi per ospitare il deposito unico nazionale per le scorie nucleari e la risposta positiva di Trino Vercellese ci fa capire che stiamo andando nella giusta direzione. Per garantire, d'altronde, la sicurezza energetica del Paese, conciliandola con la decarbonizzazione, non possiamo affidarci solamente al sole e al vento. Ma dobbiamo necessariamente investire nella ricerca proprio sul nucleare, che è fonte sicura e sostenibile, e creare - usando ancora le parole del vice ministro Gava - un'alleanza industriale per i piccoli reattori, sviluppando una filiera energetica europea. Accanto a questa fondamentale innovazione, ne abbiamo poi introdotte altre e precisamente misure sulle risorse geotermiche, per cui le Regioni potranno chiedere ai concessionari la predisposizione di un piano di investimenti pluriennale in cui siano contemplati anche gli interventi di manutenzione miglioramento tecnologico; interventi per la salvaguardia dell'ambiente e interventi per aumentare l'occupazione; estendiamo gli incentivi per gli impianti alimentati da bioliquido da biomasse, introduciamo norme per la realizzazione dei rigassificatori, in particolare a Porto Empedocle e Gioia Tauro, e istituiamo il fondo per la realizzazione di impianti rinnovabili nelle aree idonee, sostenendo le Regioni nel rapido raggiungimento degli obiettivi territoriali di diffusione di queste energie. Inoltre, tengo a sottolineare che proprio la Lega ha contribuito in modo determinante al miglioramento di questo provvedimento, perché proprio grazie a un emendamento del mio Gruppo sono state eliminate le tasse sulle rinnovabili, cioè il contributo annuo che era stato previsto a carico dei produttori di energia verde. Sono state poi introdotte ulteriori semplificazioni amministrative, sempre con un emendamento della Lega, come per la realizzazione di centrali termoelettriche e di impianti fotovoltaici per favorire sempre più la diffusione dell'energia *green*. Insomma, quello che stiamo per varare è un provvedimento che rende l'Italia sempre più autonoma e avanzata anche dal punto di vista energetico, mantenendo salda la propria competitività internazionale, ma con un sempre maggiore uso di energia rinnovabile e, quindi, con una sempre maggiore sensibilità verso il rispetto dell'ambiente. Basti pensare alle ulteriori misure innovative che riguardano la creazione di un polo strategico nazionale per l'eolico *offshore*, che avrà sede in due porti del Sud attraverso la realizzazione di apposite piattaforme galleggianti, e ancora alle altre misure sulla sperimentazione di nuove tecnologie per catturare e stoccare la CO2, che consentiranno di abbattere le emissioni industriali senza dover intaccare la produzione. Questo è un provvedimento, in sostanza, che forse affronta per la prima volta con visione una materia fondamentale per un qualunque Stato che voglia definirsi moderno e che per la prima volta davvero dà all'Italia i mezzi per mezzi per potersi sganciare dagli approvvigionamenti energetici esteri, per affermare sempre più la sua forza nel panorama internazionale, senza ridurre la produzione industriale o viceversa far passi indietro verso il carbone - come forse vorrebbero dall'altro lato del banco e come sta facendo, ad esempio, la

vengono dati nuovi sostegni per la ricostruzione e insieme per la ripartenza delle industrie, cosa che a noi sta molto a cuore. Per tutti questi motivi, a nome del Gruppo Lega esprimo convintamente il voto favorevole. il Governo e la maggioranza sono entrati nel Guinness dei primati fra i Riguardo ai decreti-legge, l'Esecutivo Meloni ha imposto la fiducia per oltre 50 volte in appena due anni. È gravissimo: si continua a escludere il Parlamento su priorità nazionali, a partire dai decreti-legge, che contengono tutto, abusando della decretazione d'urgenza senza alcun limite.

In un testo che tratta una materia delicata e strategica, cioè la sicurezza energetica del Paese, il Governo ha inserito di tutto e di più, per esempio il commissariamento del ciclo dei rifiuti in Sicilia, affidando al Presidente della Regione il ruolo di Commissario. Insomma, si dimostra anche in questo caso la superficialità, la lentezza e la sciatteria amministrativa del Governo, che nello stesso decreto-legge ha provato - malissimo

il problema dei rifiuti in Sicilia, i danni delle cosiddette bombe d'acqua che hanno colpito le tre Regioni andassero discussi separatamente e affrontati con tre provvedimenti diversi, coinvolgendo il Parlamento. Invece, l'Esecutivo e la maggioranza di destra seguono due strade opposte: una cosiddetta differenziata, leghista, funzionale a spaccare il Paese, e una indifferenziata, quando occorre rimediare alla propria incapacità politica di analizzare e risolvere i problemi. Il decreto-legge in esame è privo di misure per contrastare i cambiamenti climatici e ciò conferma che il Governo non ha una politica energetica ragionata ed efficace. Inoltre, siete incoerenti rispetto alle conclusioni raggiunte alla COP28, che ha riconosciuto la necessità di una transizione profonda dai combustibili fossili. fossili. Non vengono poi considerate le micro, piccole e medie imprese, che invece meritavano, in un decreto-legge come questo, misure concrete per affrontare la transizione energetica come opportunità di sviluppo e crescita.

Non doveva iniziare già dallo scorso luglio una campagna mirata? A oltre sei mesi da allora, quella campagna non esiste e non può contare su risorse efficienti. Questa occasione poteva essere utilizzata, ma ancora una volta l'avete persa, perché non avete voluto compiere una scelta di politica industriale attenta e tangibile sul problema dell'energia, che le aziende vivono con enorme ansia per il loro futuro. Peraltro, grazie alla tenacia delle opposizioni, l'Esecutivo ha evitato, per la verità con un lavoro importante soprattutto alla Camera dei deputati, l'ennesimo errore imperdonabile, perché nel provvedimento avevate tassato i nuovi impianti rinnovabili con 10 euro al kilowatt per i primi tre anni. Al riguardo siete stati bloccati e siete stati costretti a tornare indietro dopo la reprimenda delle opposizioni e degli operatori. Non è tutto: nel decreto-legge in esame prevedete che le nuove trivellazioni per la ricerca di gas avvengano anche in aree già vietate per ragioni ambientali e di sicurezza. Per di più, riguardo all'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, il provvedimento rischia di buttare letteralmente a mare tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, perché introduce le autocandidature dei Comuni perfino in aree ritenute fino ad ora inidonee per motivi

C'era bisogno di un provvedimento a parte, come vi direbbe chiunque - e mi riferisco al Governo - ma a voi non importa del buon senso: vi interessano gli *slogan*, gli *spot* e il fumo mediatico. Difatti, non avete accettato nessuna delle proposte delle opposizioni relative agli aiuti per gli alluvionati, come quelle del Partito Democratico riguardo all'Emilia-Romagna, che contemplavano risorse, puntualmente individuate, per indennizzare le famiglie rispetto ai danni subiti dai loro beni mobili. Inoltre, non è stato possibile discutere e approvare le proposte finalizzate al credito d'imposta per le imprese e per la proroga del pagamento dei mutui con Cassa depositi e prestiti per gli investimenti pubblici da parte dei Comuni alluvionati. Avete detto di no anche ai sostegni all'agricoltura, chiudendo gli occhi su tutto quello che sta succedendo nel Paese con gli agricoltori e girandovi dall'altra parte. Mentre si sta per approvare un decreto-legge in cui si sarebbero potute inserire misure che avrebbero dato immediate risposte a quanto sta avvenendo nel Paese, vi siete girati dall'altra parte. Avete respinto tutte le proposte finalizzate a favorire l'impiego delle risorse del PNRR da parte dei Comuni interessati, per i quali avevamo previsto idonei strumenti anche di personale. Analogo comportamento avete avuto sulle proposte di fondi per la ricostruzione e per i finanziamenti agevolati. Per quanto riguarda la Toscana, avete detto di no alle nostre proposte per il sostegno agli investimenti privati e l'accesso alla liquidità da parte delle imprese danneggiate dall'alluvione. Peraltro, avete escluso l'ulteriore sospensione dei termini di versamento dei tributi, così come dei contributi previdenziali e assistenziali. Per completare l'opera, non avete accolto la proposta che noi avevamo fatto di 200 milioni per l'alluvione nelle Marche, per garantire il ristoro integrale dei danni subiti. sul tema dell'energia non c'è in questo decreto-legge alcuna strategia. Non avete messo un centesimo sul Fondo per il clima, che era stato già decurtato di 280 milioni. Non avete previsto poi i termini delle compensazioni locali per le trivellazioni, alla faccia dell'autonomia differenziata che amate sbandierare quando vi fa comodo. Proprio sull'autonomia, a riprova della schizofrenia politica del Governo e delle vostre bugie sull'autonomia differenziata, avete detto no a una proposta che abbiamo fatto, che avrebbe permesso alle Regioni di avere l'ultima parola sulla scelta delle aree idonee alla ricerca e allo sfruttamento della geotermia. Sempre per il suo tramite, signor Presidente, mi rivolgo alla senatrice della Lega che è intervenuta prima.

e le aree da usare per la geotermia. In questo decreto poi non viene dato alcun incentivo alle imprese, specie a quelle che utilizzano le energie rinnovabili. ancora una volta avete forzato la mano e avete imposto i vostri tempi e il vostro consueto disordine; ancora una volta, avete mortificato questo Parlamento. Considerato il ruolo strategico della sicurezza nazionale e vista l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici e la necessità che in materia di energia l'Italia abbia una politica lungimirante, come Partito Democratico avevamo presentato molte proposte valide e fattibili, nonostante la fretta imposta dal Governo, appoggiato da una maggioranza silente, supina e remissiva. Voglio ricordare che avevamo chiesto di valorizzare le imprese agricole impegnate nella produzione di energia di fonti rinnovabili; si tratta di imprese che concorrono in maniera significativa al progetto di transizione ecologica ed energetica, dunque al contrasto dei cambiamenti climatici. Avevamo anche chiesto di inserire nel provvedimento nel provvedimento la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale. Anche al riguardo, siete stati sordi, ciechi e chiusi. chiusi. Non ci resta che farvi i complimenti per l'allergia che avete al confronto parlamentare, per la vostra sfacciataggine politica e per la vostra arte dell'arrangiarvi. per la vostra mancanza di visione e prospettiva e per la vostra insensibilità rispetto alle condizioni delle imprese, delle famiglie, degli alluvionati e dei consumatori. Come sempre, avete voluto agire da soli e vi siete arroccati sulle vostre posizioni, dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, la vostra avversione per il confronto, la democrazia e i bisogni veri del Paese. Dunque, esaminato nel merito e nel metodo, questo vostro decreto-legge non garantisce affatto la sicurezza energetica del Paese. È invece l'ennesimo, inutile provvedimento *spot*, che fa male all'Italia, fa male agli italiani, fa male ai consumatori, fa male ai cittadini e fa male ai portatori di interesse; insomma, non risponde alle esigenze di questo Paese. Per questo, in maniera convinta, voteremo contro sicuramente alla fiducia a questo Governo, perché non la merita, ma anche nel merito del provvedimento siamo per un voto nettamente contrario.

per la sicurezza energetica del Paese, per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e gas e per favorire la ricostruzione delle attività produttive nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Su quest'ultimo punto, ovvero sui provvedimenti per i territori delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, ritengo ci sia poco da dire non perché non siano importanti, ma perché condivido quanto detto ieri dalla collega Farolfi che, rispondendo alle accuse della minoranza, ha dettagliato quanto fatto in favore dei territori citati, smentendo qualsiasi critica, chiaramente strumentale. Il Governo Meloni ha assunto impegni, come doveva, e anche con quest'ultimo provvedimento mantiene la parola data. Non esistono, come qualcuno ha voluto insinuare, territori di serie A o di serie B, a seconda di chi li governa. Non più di pochi secondi vorrei dedicare all'ulteriore trovata delle opposizioni quando citano il titolo di un quotidiano, secondo il quale con il Piano Mattei verrebbero sottratte risorse al fondo per il clima. Basta leggere l'articolo 13 del decreto-legge, che invece rifinanzia il fondo con ulteriori 200 milioni di euro per il 2024, portandolo a 1,04 miliardi di euro. inoltre difficile commentare le corbellerie del senatore Trevisi, del MoVimento 5 Stelle, che dimostra di non conoscere assolutamente la situazione africana, richiamando parole ad effetto come il colonialismo; banalità, pur di parlare. Vorrei invece soffermandomi sulla parte più corposa del provvedimento, le norme con le quali si incentiva la transizione energetica del Paese, senza dimenticare, al contempo, il tessuto produttivo ed economico italiano, questa, che richiede attenzione e tempestività di decisioni e quindi necessita delle dovute misure, adottate anche con provvedimenti d'urgenza, che l'opposizione critica dimostrando troppo facilmente di dimenticare il recente passato. La situazione energetica è sicuramente un settore in cui dobbiamo accelerare e fare più di quanto fatto in passato. Non penso quindi che lo strumento del decreto-legge sia in questo caso inappropriato non ritengo che questo Governo ne abusi, anche considerando i dati degli ultimi Governi, che ci consegnano una media di due decreti-legge pubblicati al mese. Senza contare, senatore Irto, il corposo numero di provvedimenti adottati durante i Governi Conte I e Conte II senza modifiche da parte di un ramo del Parlamento; solo in nove occasioni si è resa necessaria la famosa navetta. Questo per dire ai colleghi dell'opposizione che sarebbe il caso di abbandonare certi atteggiamenti da censori, che non si possono permettere di entrare nel merito delle questioni, se vogliono davvero essere responsabili. Ne gioverebbe la qualità del dibattito politico. Purtroppo in quest'Aula, ma anche al di fuori, assistiamo a un tale sterile tentativo di andare contro la maggioranza, che si finisce per dire di tutto: che siamo contro la decarbonizzazione, che vogliamo alimentare le disuguaglianze ambientali, sociali ed economiche e altre assurdità dello stesso genere. Se le opposizioni abbandonassero per un attimo l'ipocrisia che colora la contrapposizione politica forzata, si renderebbero conto che questo provvedimento è concreto e va verso una seria transizione energetica, rimanendo con i piedi per terra. L'accusa più assurda, ascoltata di continuo, è che saremmo contro la decarbonizzazione: detto da chi oggi critica i rigassificatori, ma ieri appoggiava il Governo Draghi, che ha definito quello di Piombino essenziale per la sicurezza energetica nazionale, è ridicolo. *(Applausi)*. È ancora più ridicolo se si pensa che, nonostante le prese di posizione dei partiti che lo sostenevano, MoVimento 5 Stelle incluso, Draghi non è certo caduto per il suo sostegno al rigassificatore. La collega, senatrice Naturale, oggi è andata oltre e ci ha detto di essere anche contro l'eolico *offshore* - aggiungo io - con buona pace degli ambientalisti, ma anche del suo stesso collega, senatore Trevisi, che nel suo intervento ha speso

Personalmente, avendo bene a mente gli impegni assunti dall'Italia, ritengo che sia ora di smetterla con le affermazioni ideologiche e di bandiera che non fanno bene al futuro del nostro Paese. Per fare ciò bisogna partire dalla realtà dei fatti. Innanzitutto, è necessario essere coscienti del fatto che neutralità climatica significa non zero emissioni, ma che quelle prodotte devono essere compensate da quelle assorbite. Questo significa: trovare un equilibrio un equilibrio che, passo dopo passo, l'Italia vuole raggiungere. Basti pensare, al contrario degli *slogan* dell'opposizione, che tra il 2021 e il 2023 i nuovi impianti di energia rinnovabili sono cresciuti di oltre il 400

a diminuire l'approvvigionamento di gas dall'estero, né l'uso dello stesso gas) che non possiamo ridurre il portafoglio dell'energia al solo eolico e fotovoltaico. Semplicemente non si può, perché l'attuale tecnologia non lo permette e - soprattutto - non si può fare senza assicurare una transizione sostenibile per tutti. Questo non lo dice il Governo Meloni, ma lo dicono la Commissione europea, il Parlamento europeo e chiunque si occupi di energia. il mondo intero, tranne l'opposizione, il cui unico fine è quello di menare il can per l'aia. Ricordo a me stesso - e sarebbe il caso che le opposizioni facessero attenzione - che la tassonomia europea, ovvero il sistema di classificazione che stabilisce i requisiti delle attività economiche ecosostenibili e che serve a orientare gli investimenti per accelerare la transizione ecologica degli Stati membri, contempla nel *mix* energetico anche gas e nucleare, oltre alle classiche forme di energia prodotta dalle fonti rinnovabili. Si è infatti finalmente compreso che la transizione energetica non è un monolite di pietra impermeabile a tutti gli altri settori della vita sociale ed economica. Non si può parlare di transizione energetica senza tener conto della sicurezza energetica nazionale e della sostenibilità economica delle scelte. Non si può pensare di eliminare il gas (che nel *mix* energetico pesa per circa il 47 per cento) dall'oggi al domani senza mettere in conto il collasso del sistema Italia. Qualcuno dirà che l'Accordo di Parigi risale al 2015, ben otto anni fa, ma ricordo a tutti noi che in questi anni hanno governato altri e noi, responsabilmente, stiamo recuperando quello che non è stato fatto prima. L'Italia è il secondo Paese in Europa per industria manifatturiera che, come si sa, è costituita da settori fortemente energivori: ceramica, vetro e industria chimica, metallurgica e dell'acciaio. Cosa dovrebbero fare queste aziende mentre si sviluppa la produzione dell'idrogeno verde? Cosa dovrebbero fare le aziende che ancora non hanno le tecnologie per elettrificare i processi produttivi? Chiudere? Ecco perché esame va verso una transizione energetica sostenibile e concreta, priva di ideologie. Ad esempio, da un lato prevede misure per promuovere l'autoproduzione di energia, incentivi a ospitare impianti a fonti rinnovabili, semplificazioni in materia di procedimenti e incentivi agli impianti alimentati da biomassa e biometano. Dall'altro lato, il provvedimento non dimentica ad esempio che ci sono settori ancora alimentati da fonti fossili che producono CO2 che difficilmente, dall'oggi al domani, possono diventare totalmente a impatto zero e lo fa colmando alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio di CO2 (articolo 7). Questo si chiama affrontare le questioni a 360 gradi, altro che essere contro la decarbonizzazione. *(Applausi)*. Poi, tra le tante parole dell'opposizione, mi fanno sorridere quelle con le quali ci dicono che vogliamo alimentare la disuguaglianza ambientale e al contempo criticano la scelta del nostro Governo di dare la possibilità alle comunità di avanzare le proprie candidature per essere sedi del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Innanzitutto, a differenza delle accuse mosse, non si danneggia alcun territorio, né si rendono idonei territori che sono invece inidonei. La norma prevede esplicitamente - e lo sottolineo - non solo strategica (VAS), ma anche una successiva valutazione di idoneità del sito da parte della Sogin rispetto all'autocandidatura. La differenza tra noi e voi è che mentre voi criticate questa norma, per noi è l'espressione del rispetto dell'autodeterminazione delle nostre comunità, Grazie, lì, le opposizioni hanno fatto a gara a muovere accuse di immobilismo contro il Governo Meloni. I fatti dimostrano il contrario, tanto che oggi, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale approvato da Bruxelles, arrivano le regole e soprattutto le risorse. le risorse. Ogni cosa che si mette in campo per le opposizioni non va bene, poi però arrivano gli effetti positivi dei provvedimenti e si deve tacere. Anche oggi si ripete lo stesso spartito. In conclusione, il provvedimento in esame rappresenta un altro passo avanti per portare a compimento la strategia energetica di questo Governo e di questa maggioranza al fine di garantire all'Italia la sicurezza energetica. È un altro passo in avanti verso la neutralità climatica, senza dimenticare la sostenibilità economica e sociale senza la quale non sarebbe possibile realizzare nulla. Per questi motivi, non posso che annunciare con convinzione il voto favorevole e la conferma della fiducia del Gruppo Fratelli d'Italia.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

chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro chiusa la votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge

intervengo per sottoporre ai colleghi un tema che noi riteniamo increscioso, per il quale abbiamo

che mette i Gruppi di opposizione in questa condizione). Vorrei, signora Presidente, sottoporre alla sua attenzione

durante la discussione dell'emendamento 13.0.1 (che - per capirci - faceva riferimento alla proposta di salario minimo nella legge di delegazione europea, quindi nella legge comunitaria),

Il senatore Lorefice e la senatrice Malpezzi sono intervenuti subito dopo per sottolineare come questo non fosse né corretto, né rispettoso. La sottosegretaria Siracusano ha esplicitato, successivamente a questa forzatura, la sua motivazione e il parere.

Presidente Malan, presidente Gasparri (non vedo il presidente Romeo), può accadere che in quel momento la maggioranza non sia compatta, non sia presente o non la pensi in quel modo, non per questo un Presidente di Commissione può permettersi di non far rispettare le regole o di accelerare all'improvviso il processo di voto, stabilendo che si vota mentre non è stata fatta la dichiarazione di voto.

dai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari di opposizione. Per questo chiediamo che, a norma dell'articolo 18, comma 3-*bis*, del Regolamento del Senato venga convocata immediatamente la Giunta per il Regolamento, perché questo è per noi inaccettabile.

tutelare tutti noi, maggioranza e opposizione, e non solo la maggioranza. Signora Presidente, aggiungo un tema che abbiamo posto all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo di ieri. Da sei mesi aspettiamo su un affare assegnato il ministro Fitto. Oggi leggiamo sulla stampa che il ministro Fitto e il ministro Giorgetti continuano a litigare sul PNRR, tanto che il Consiglio dei ministri non ha deliberato il via libera su quei 19 miliardi attesi dai territori, dagli enti locali e dalle Regioni, su cui si stanno scaricando tutti i ritardi che il Governo sta sommando in questo momento. momento. Abbiamo più volte detto al Governo che il tema non è ottenere la rata (forse la rata la otterrete, soprattutto se barate e non dite la verità a Bruxelles); il problema è se le risorse ottenute da quelle rate arriveranno sui territori. Non solo non stanno arrivando, ma ci ritroviamo centinaia e centinaia di Comuni e molte Regioni che hanno appaltato le gare e ora non hanno le risorse. Il Governo si sta già inventando un tema che non ci piace, cioè ossia quello della burocrazia delle Regioni e degli enti locali che rallenterebbe i lavori. No, signora Presidente, non c'è nessuna burocrazia dei Comuni e delle Regioni; c'è la burocrazia del Governo e c'è un Governo che continua a litigare sulle finalità ed il tema che più ci sta a cuore. Per questo motivo, le chiedo, a nome del Partito Democratico (e immagino di interpretare il sentimento anche di tutti gli altri Gruppi di opposizione su questo tema), di sollecitare il ministro Ciriani a darci una data in cui il ministro Fitto, non certo non rispondeva a una curiosità delle opposizioni, ma semplicemente rispetta Palazzo Madama, viene qui,

principale che ha posto il presidente Boccia, parlando a nome di tutte le opposizioni che hanno firmato la lettera a cui si è

Parlo evidentemente senza aver letto la lettera e le comunicazioni scritte fatte dal presidente Boccia e dagli altri colleghi dell'opposizione,

fattualmente risposto con una mia dichiarazione, così come hanno anche risposto alcuni altri colleghi della maggioranza a seguito di questa diversità di interpretazione di come siano andate le cose. Premetto che confido sul resoconto puntuale, non di verbalizzazione testuale, ma di sintesi, di quello che è stato il dibattito e del punto che è stato presentato soprattutto dal senatore Filippo Sensi. È avvenuto che nella discussione degli emendamenti di un articolo, al quale erano riferiti una serie di emendamenti, si è

emendamento; ai sensi del Regolamento, chi illustra può presentare anche gli altri emendamenti sullo stesso articolo che ha firmato, essendo titolare della proposta di emendamento. è poi passati alla valutazione del relatore e del Governo e, quindi, alle dichiarazioni di voto. Questo è avvenuto puntualmente - sottolineo puntualmente - nella votazione incriminata dal senatore Sensi - mi permetta di usare questo termine - e ritenuta illegittima perché non erano ancora stati ripensati alcune posizioni e commenti

eletto da un certo numero di miei cittadini che mi hanno portato in questa Aula per esprimere il mio parere e il mio voto in ogni situazione nella quale questo voto ritengo debba essere proposto. Non accetto intimidazioni neanche di natura politica, con dichiarazioni, presenze, blocco dei lavori o falsità che vengono esposte sull'ordine dei lavori che è stato da me condotto, con il parere anche positivo della maggioranza, ma non solo della maggioranza, di chi era presente. Non accetto intimidazioni di sorta o bavagli, come amate dire e come amano dire i colleghi dell'opposizione

alla mia indipendenza di giustizia e alla mia volontà di essere *super partes* e di favorire costantemente un avvicinamento di posizioni

di un'interlocuzione fra relatore e portavoci dell'opposizione per la presentazione di un emendamento o, in alternativa, di un ordine del giorno. Questa è la versione dei fatti, signora Presidente. Sono disponibile per chiarirne i dettagli, i passaggi, le cose dette e le frasi - mi consenta - ingiuriose nei miei confronti, che non tollero, espresse in quell'occasione.

da tutti i Capigruppo dell'opposizione. Evidentemente c'è una questione, che è stata circostanziata sia da chi ha proposto la lettera, sia da lei, e anche un insieme di valutazioni che, come dicevo, non potranno che essere riferite al Presidente, per le opportune valutazioni sulla convocazione della Giunta per il Regolamento e non solo. Sicuramente in quest'Aula non sono state pronunciate frasi ingiuriose, perché non lo avrei ovviamente consentito. Come avevo già detto, la questione non è oggetto di dibattito ulteriore. Hanno parlato un esponente dell'opposizione, a nome di tutti, e un esponente della maggioranza direttamente chiamato in causa, come il Presidente della Commissione.

Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, Governo, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 924, di iniziativa del Governo collegato alla legge di bilancio, approvato dalla 7a Commissione permanente lo scorso 21 dicembre. La Commissione, all'esito dell'esame in sede referente del testo risultante a seguito dello stralcio delle disposizioni in materia di valutazione del comportamento degli studenti, è pervenuta alla definizione di un testo senz'altro arricchito, con l'accoglimento di diversi emendamenti avanzati dai Gruppi sia di maggioranza, sia di opposizione, a conferma di un clima di sereno confronto favorito dal presidente Marti, a cui va il mio personale ringraziamento. Quello in esame è un testo in grado di porsi come valido strumento normativo per rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle inderogabili richieste di qualificazione specialistica provenienti dal settore imprenditoriale. Signor Presidente, oggi in Italia c'è una reale difficoltà di reperire figure professionali specializzate, figure nuove che sono richieste dal mercato del lavoro. Dall'ultima indagine di Unioncamere e ANPAL risulta che, su 508.000 assunzioni programmate dalle nostre imprese, purtroppo 205.000 pagano lo scotto di non avere candidati formati oppure con una formazione non adeguata. Questo ci dice tutto. È evidente che la scuola, in questo momento, è distante, in termini di competenze e in termini di formazione, rispetto a quello che chiede oggi sempre più il mondo del lavoro. Il disegno di legge, composto da quattro articoli, reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e attuata dagli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, in tal modo contribuendo a quello che è il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione. L'istituzione della filiera intende, quindi, realizzare l'interconnessione che deve necessariamente sussistere tra l'offerta formativa

alle esigenze economico sociali e soprattutto alle caratteristiche dei territori. Tali contenuti consentono, quindi, ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata, più formata, anche sotto un profilo tecnico e pratico. L'articolo 1, mediante l'inserimento di un apposito articolo, il 25-*bis*, nel decreto-legge n. 144 del 2022, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, nella quale sono ricompresi: i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che saranno attivati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori, ITS Academy, di cui alla legge n. 99 del 2022; i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; infine, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio del 2008. Come ho già detto, il provvedimento in esame, nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale. Con apposite disposizioni, viene pertanto disciplinato il ruolo delle Regioni nell'ambito della nuova filiera. In particolare, si stabilisce che, ferme restando le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, le Regioni possono aderire alla filiera mediante la stipula, con gli uffici scolastici regionali, di accordi funzionali alle esigenze specifiche dei territori e finalizzati ad ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali. I suddetti accordi possono anche prevedere le istituzioni di reti, denominate *campus*, in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte. Al comma 6 del nuovo articolo 25-*bis* sono espressamente individuati i contenuti dei predetti accordi e dei percorsi sperimentali, che saranno attivati ai sensi del comma 2: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, assolutamente imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, al fine di supportare l'importante criticità dovuta al ritardo con il quale i nostri giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari. Vi è poi il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione, nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche. Sono altresì individuati i contenuti facoltativi dei medesimi accordi, tra i quali l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti e delle attività formative programmate in lingua straniera; la promozione di accordi di partenariato, la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzate all'interno dei percorsi formativi della nuova filiera, e il trasferimento tecnologico verso le imprese. Sono poi disciplinate le modalità di accesso agli ITS Academy da parte dei soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale. L'accesso diretto agli ITS Academy da parte dei soggetti che hanno concluso il percorso quadriennale costituisce uno degli aspetti fondamentali e soprattutto innovativi del provvedimento in esame e la vera sfida di questo provvedimento. È infine disciplinata la possibilità per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di Invalsi, di sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale di competenza, senza dover previamente sostenere l'esame preliminare. L'articolo 2 provvede all'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione del merito, di una struttura tecnica di livello dirigenziale a cui è affidata un'importante missione, quella di promuovere la filiera formativa, tecnologica e professionale. Alla struttura tecnica sono attribuite in particolare le funzioni di promuovere le sinergie tra la filiera formativa, tecnica, tecnologica e professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico; di ampliare la progettazione dei percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese, di favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Invalsi. L'articolo 3 disciplina l'istituzione, presso la suddetta struttura tecnica, di un Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa, tecnologica e professionale, al quale è attribuito il compito di proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa, formativa, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Infine, l'articolo 4 istituisce il Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024

colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che discutiamo oggi avrebbe l'obiettivo di riorganizzare il percorso formativo dell'istruzione secondaria professionale di secondo livello che coinvolge gli istituti tecnici, gli istituti professionali e la formazione regionale. Questo è un provvedimento che giunge in Aula ampiamente emendato. E colgo l'occasione per suo tramite, signor Presidente, per ringraziare sia il Presidente della Commissione, sia la relatrice Bucalo che, nonostante fossero incalzati dal Governo, hanno permesso un'ampia discussione e anche l'accettazione di numerosi emendamenti. Tuttavia, ci sono ancora, per quello che ci riguarda, alcuni aspetti critici che colgo qui l'occasione per evidenziare e non posso fare a meno di discutere di che cosa cambia rispetto alla situazione attuale, ovvero il *curriculum* degli studi

- l'incremento delle ore pratiche e di laboratorio; il coinvolgimento nella didattica e nella formazione di personale che viene dal mondo imprenditoriale e dal mondo del lavoro del territorio in cui l'istituto professionale ha sede; l'autonomia dei singoli istituti a progettare percorsi per competenze trasversali e orientamento. Particolare enfasi viene posta sull'apprendimento della lingua inglese e sulla valorizzazione della proprietà intellettuale. Trattandosi però di giovani, pieni di entusiasmo e di inesperienza nel momento in cui affrontano il lavoro, penso che manchi una formazione sulla sicurezza del lavoro. In Italia, ogni anno muoiono più di 1.000 persone per incidenti sul lavoro e per questi giovani che indirizziamo al lavoro così presto forse una formazione di questo tipo sarebbe auspicabile. il modello organizzativo cambia, come è stato evidenziato dalla relatrice. Cambiano le modalità di accesso all'ITS Academy; cambia il requisito per l'esame di Stato per alcune categorie e poi c'è la formazione delle reti didattiche che coinvolge l'ITS Academy, le università, le industrie e - come è stato detto - le Regioni. Ci sono sicuramente degli aspetti estremamente positivi in questa impostazione, ma non si può fare a meno di sottolineare che è un indirizzo formativo strettamente ancorato al territorio, chiaramente per sfruttare le competenze e le opportunità che il territorio può offrire. È chiaro, però, che questo avviene a spese di una frammentazione della formazione e anche, forse, in assenza di una attività e di un'offerta formativa comune con *standard* uguali su tutto il territorio nazionale, perlomeno su alcuni aspetti. Tutto questo ha una ricaduta sulle opportunità dei nostri studenti. È chiaro, a questo punto, che uno studente, che inizia un percorso professionale al Sud e in un'area poco industrializzata e con poche offerte, ha un un percorso formativo completamente diverso da quello di uno che invece magari ha la fortuna di trovarsi nel distretto industriale Monza-Brianza o Treviso-Vicenza-Padova. Ho presentato

nelle strutture che evidentemente possono offrire più opportunità di formazione e di inserimento. Spero che questo ordine del giorno venga preso sul serio, perché effettivamente può fare la differenza per diminuire le disuguaglianze tra Nord e Sud e tra aree sviluppate e aree poco sviluppate. poco sviluppate. La polarizzazione della formazione ha anche altre conseguenze che interessano tutti gli studenti e che non possono essere ignorate. La focalizzazione del *curriculum* verso l'inserimento degli studenti in attività produttive sul territorio avviene a spese di competenze trasversali e trasferibili. E sono queste competenze, trasversali e trasferibili, che possono essere utilizzate indipendentemente dal lavoro e possono aiutare gli studenti a cambiare lavoro in un momento in cui la nobiltà caratterizza così tanto il mondo lavorativo.

per accelerare l'inserimento nel mondo del lavoro. L'istruzione, anche se professionale, deve avere l'obiettivo di formare dei cittadini, non utili ingranaggi a un processo produttivo. Una persona alla quale la scuola abbia negato determinate competenze trasversali e trasferibili avrà difficoltà a cambiare lavoro, se questo accade o se si trova in questa condizione. Questa è una persona vulnerabile sul piano dei rapporti di lavoro, quindi sicuramente meno libera, e questo non ci piace.

c'è una differenza fondamentale tra un esperimento e un cambiamento senza base razionale. Sono tre gli elementi: il disegno sperimentale, gli indicatori misurabili e il punto di arrivo. arrivo. Questo disegno di legge, però, giunge in Aula senza queste caratteristiche, per cui non capisco cosa sperimentiamo, cioè cosa misuriamo. A questo punto questo cambiamento può avere tre effetti (neutro, negativo o positivo) e a me piacerebbe sapere

che introduciamo un cambiamento senza una *ratio*, senza un disegno sperimentale. Badate bene che se è sperimentale, questa misura ha un impatto sulle vite delle persone e, quindi, ha un aspetto etico. Quando introduciamo una cosa sperimentale, dobbiamo considerare se stiamo facendo del danno, calcolare il rischio, perché alla fine abbiamo a che fare con delle persone.

che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli ITS Academy, dai percorsi di istruzione e formazione professionale e da quelli di istruzione e formazione tecnica superiore. Inoltre, è stato previsto che anche le Regioni possano aderire alla filiera formativa tecnologica. Ho appreso a mezzo stampa le parole trionfanti della ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, per cui questo provvedimento consentirà ai giovani e alle famiglie che scelgono questo percorso di raggiungere tutti i più alti livelli dei titoli terziari e post terziari: diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, lauree, dottorati in apprendistato duale di terzo livello. Mi chiedo se il Governo, o quando meno la maggioranza, abbia mai prestato ascolto alle parole espresse dalle parti sociali, che hanno bocciato *in toto* questo provvedimento, esprimendo un giudizio fortemente negativo, atteso il generale impoverimento dell'impianto didattico che si viene a realizzare. Lo ribadiscono, ad esempio, a gran voce CGIL e FLC-CGIL, che esprimono grandissima preoccupazione. Onestamente, non si comprende tutta questa fretta, tutta l'attenzione e tutto l'interesse nel portare avanti così velocemente tale provvedimento; o meglio, si intuisce leggendo la relazione illustrativa, dove scorgiamo l'evidente *assist* che questa riforma intende offrire agli enti privati e alle aziende, che sembra si sostituiscano alla definizione dei programmi educativi, dettando addirittura i tempi dei percorsi formativi. È chiaro il tentativo, sempre più spinto da parte di questo Governo, di privatizzare tutto, dalla sanità alla scuola, come emerge dalla lettura del testo. Tuttavia, le priorità sono altre: penso ad esempio alla necessità di garantire il tempo pieno nelle scuole, soprattutto nelle aree più disagiate del Paese; un'iniziativa che offrirebbe agli studenti maggiore opportunità di apprendimento, contribuendo a ridurre le disuguaglianze educative e a fornire un importante supporto sociale ed emotivo, contribuendo anche a ridurre il rischio di coinvolgimento in attività criminali. Ma si tratta di una scelta che viene da lontano, giacché già dal tempo degli anni Settanta e Ottanta si è deliberato in maniera scientifica lo smantellamento delle scuole di secondo grado a tempo pieno, che faticosamente i politici oculati degli anni Sessanta avevano attuato. Se, come recita il testo, l'organico potrà essere integrato con contratti di insegnamento stipulati con esperti provenienti dal mondo delle imprese, chiederei alla ministra Calderone se è sicura che gli insegnanti abbiano letto questo provvedimento. In sintesi, state legittimando di mettere sotto contratto *manager* e imprenditori e lasciare a casa gli insegnanti, che già nascono tra contratti precari e supplenze *(Applausi)*, in spazi logistici obsoleti e che spesso non rispondono ai requisiti minimi di agibilità. Lo diciamo senza giri di parole, accogliendo le istanze provenienti dagli auditi: istituire relazioni stabili di coprogettazione dell'offerta formativa con le aziende e le realtà produttive del territorio rappresenta un rischio enorme soprattutto per l'autonomia didattica. Si tratta, in sintesi, dell'ennesimo colpo di grazia che state dando al mondo della scuola, al personale ATA, al corpo docenti e soprattutto alle nostre figlie e ai nostri figli. State svendendo la scuola al privato, abbreviando i percorsi didattici e anticipando le esperienze lavorative. Ma soprattutto state impoverendo il concetto stesso di istruzione che, per noi, rimane legato a una comunità educante, ignorando le vere criticità che provengono dal mondo della scuola. Penso alla sicurezza dei nostri figli, laddove, dal ventesimo rapporto Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola redatto da Cittadinanzattiva, emerge che il 58 per cento degli istituti scolastici italiani non ha il certificato di agibilità statica e di prevenzione incendi, mentre oltre il 40 per cento è privo del collaudo statico, anche a fronte undici Regioni che presentano un elevato rischio sismico. Queste sono solo alcune fra le priorità su cui si dovrebbe intervenire. Il MoVimento 5 Stelle ha dato il massimo per arginare le numerose criticità di questa riforma, presentando moltissimi emendamenti che avete respinto al mittente, temendo qualche corto circuito rispetto al vostro piano di privatizzare gli ITS. Nonostante la maggioranza avesse remato in direzione diametralmente opposta rispetto al buon senso, non ha potuto però non approvare un mio emendamento - e di questo vi ringrazio - che recava l'obiettivo di aiutare gli studenti disabili. modo, grazie a una proposta emendativa del MoVimento 5 Stelle a mia prima firma, riusciremo quantomeno a sostenere, durante il loro inserimento nei contesti lavorativi, i soggetti più fragili. È cruciale che istituzioni educative, organizzazioni e comunità si impegnino a promuovere una cultura dell'accettazione, dell'accoglienza, dell'empatia e del sostegno reciproco e, cioè della condivisione. Pertanto, occorre lavorare insieme per abbattere le barriere sia fisiche che sociali che impediscono alle studentesse e agli studenti disabili di partecipare pienamente alla vita accademica e professionale, a sperimentare il comune vivere delle difficoltà che la vita presenta nel quotidiano. Onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo a dibattere di una scatola vuota, dell'ennesimo provvedimento propagandistico che portate a casa solo per tornaconto politico elettorale e che ha l'esclusivo obiettivo di rispondere agli interessi di un sistema scolastico privato, fortemente supportato dalle *lobby*. Non è questo il modo di trattare la nostra scuola, il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno. Il sigillo di questa riforma è il marchio della disuguaglianza ed espressione propria di un Governo che è già passato alla storia come il pallido custode dell'ingiustizia e dell'abbandono di 60 milioni di italiani. Tuttavia, non voglio concludere questo mio intervento con un concetto così triste, una presa d'atto di un provvedimento, l'Atto Senato 924, del tutto disancorato da quanto si sarebbe potuto fare. L'auspicio è che questo Governo, presieduto da una donna, Giorgia Meloni, possa ravvedersi, osservare con più attenzione i bisogni dei giovani e della società, e possa attuare quei cambiamenti nel mondo scolastico, anche per ridurre l'abbandono, la mortalità scolastica e, in sintesi, quella povertà educativa che in alcune realtà ha raggiunto proporzioni allarmanti.

qui lei oggi. Senza nulla togliere alla Sottosegretaria, trovandoci di fronte alla discussione generale di un provvedimento che è una riforma del mondo dell'istruzione, ci saremmo però aspettati la presenza del Ministro, che forse dovrebbe venire in Parlamento anche ad ascoltare quello che è il dibattito. Verrà magari per le dichiarazioni di voto, ma avrei preferito poterlo vedere anche per il dibattito. Cara Cara Sottosegretaria, ci troviamo di fronte a un'occasione mancata. Perché ci troviamo di fronte a un'occasione mancata quando affrontiamo questo provvedimento? La fretta rischia di fare i gattini ciechi. Diceva così un vecchio proverbio contadino: la gattina furiosa ha fatto i gattini ciechi. Il provvedimento nasce per provare a dare una risposta alla dispersione scolastica; provare a rendere la nostra scuola, per alcuni aspetti, anche vicina - come ricordava prima la relatrice in un passaggio - ai sistemi europei; per provare a garantire ai ragazzi una diversificazione anche di formazione a seconda delle proprie intelligenze emotive. Non tutti apprendono nello stesso modo e, proprio perché serve una scuola che risponda alle esigenze dei ragazzi, è bene che la scuola stessa si interroghi e possa anche cimentarsi in riforme. Quando però le riforme e i grandi cambiamenti vengono fatti così in fretta, io

Perché dico che ci sono dei rischi? Ce lo dicono i numeri di chi ha aderito alla sperimentazione. Vorrei sottolineare quello che il collega Crisanti prima ha detto. Noi siamo di fronte a una sperimentazione, a una riforma sperimentale o a un vero e proprio cambiamento di passo? Quando in Parlamento è arrivato questo provvedimento di riforma, ci siamo trovati subito dopo le scuole che ci chiamavano perché era arrivata una circolare che diceva loro di far partire la sperimentazione. Diceva loro cioè che il Parlamento stava discutendo,

e voi sapete, perché la scuola la frequentate - nel senso che la frequentate dai banchi del Governo, perché vi occupate delle norme che la riguardano - che c'è un termine per le iscrizioni al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, che è dovuto slittare sia per questa sperimentazione che per il liceo *made in Italy*. Italy*. Le scuole non hanno avuto neanche il tempo di poter dire che vogliono cimentarsi in questo grande cambiamento, perché nel giro di tre settimane dovevano convincere i collegi dei docenti ad aderire alla proposta e rivoluzionarsi al loro interno. Cosa è successo? Cosa ci dicono i numeri? che hanno aderito a questa sperimentazione, che ha come finalità anche quella di dare una risposta alla dispersione scolastica, di provarci, di aprire uno sguardo diverso rispetto a un settore importante come quello tecnologico-professionale, solo le scuole che erano già pronte a un'innovazione, con una grande discrepanza rispetto al resto del Paese. Pensate per esempio che la Lombardia è quella che ha avuto il numero più alto di adesioni. I numeri sono usciti l'altro giorno, li ha mandati in giro il Ministero: ci sono 176 istituzioni scolastiche che hanno deciso di partecipare alla sperimentazione, su 1.700 che avrebbero potuto Per carità, erano libere di farlo. Ma il fatto che solo 176 lo abbiano fatto, quando la finalità è così importante, come quella che voi avete delineato nella relazione della collega Bucalo, significa che qualche difficoltà nell'organizzazione c'è. La maggioranza di queste istituzioni sono in Lombardia oppure sono laddove la sperimentazione sui professionali e sull'istruzione e formazione professionale è già avanzata. che è al secondo posto rispetto a queste richieste e a queste adesioni, e l'altro la Calabria. Erano già pronte, perché stavano lavorando su una determinata filiera. Ecco che allora c'è un problema, perché il resto d'Italia fa fatica. Voi capite bene che, se fate partire una sperimentazione, che rischia di non essere sperimentazione e di andare poi a norma, perché stiamo correndo su questo provvedimento, le scuole non sono pronte ad aderire. Onde evitare che qualcuno possa pensare che io abbia pregiudizi sui quadriennali, vi dico che una delle mie figlie va in un quadriennale e fa già una sperimentazione quadriennale. È bene ricordare che si tratta di una sperimentazione che è in corso dal 2008 2008 e che è stata poi ripotenziata. Una delle mie figlie ci va. La sua scuola è una di quelle che in Lombardia ha aderito anche alla sperimentazione di filiera tecnologico-professionale. Ma è chiaro che per loro è più facile, perché hanno già un'abitudine, anche nella didattica e nella valutazione per competenze, che agevola il passaggio. Quei ragazzi forse potranno godere di uno strumento in più, ma questo non è dato a tutta Italia. Allora è lì il tema delle disuguaglianze, che non è accessibile a tutti. Devo riconoscere che il presidente Marti ha fatto uno sforzo enorme, con il suo emendamento, per mettere le risorse sui *campus*. però, dovevano essere impiegate in primo luogo per aiutare gli insegnanti a formarsi a una didattica per le competenze, che aiuta il passaggio dai cinque ai quattro anni. Se queste risorse non ci sono, le scuole faranno fatica e ancora una volta - ecco lì l'occasione mancata - una possibilità che poteva esserci, con tutta una serie di limiti che anche altri colleghi metteranno in evidenza, diventa una possibilità che verrà data a pochi. Perché avete voluto correre?

a dare una mano alle altre scuole a cimentarsi in questo. Questa poteva essere un'opportunità. Si poteva anche lavorare tutti insieme. Non faccio parte di quella Commissione, ma so che c'è stato un bel clima in 7a, per quanto anche lì un po' di corsa, senza capirne i motivi, soprattutto quando, a ridosso dell'incardinamento del provvedimento qui al Senato, il Ministro - ricordo non è presente mentre noi stiamo discutendo di questa importante riforma - aveva deciso di far partire subito la circolare. un'occasione mancata. Le innovazioni possono sempre far paura ed essere viste con uno sguardo di sospetto, anche dal mondo della scuola (posso dirlo perché provengo da quel mondo, quindi so che spesso ci sono tante paure), ma funzionano quando partono dal basso, cioè quando si riesce a far partire un coinvolgimento il più ampio possibile. Se partono gli istituti che già sono pronti a sperimentare, forse un buon servizio al mondo della scuola e soprattutto ai nostri ragazzi non lo abbiamo fatto, perché il prossimo anno scolastico partirà con sperimentazioni che non verranno attuate in tutta Italia. Vi saranno, sì, in tutte le Regioni, ma con gradazioni diverse, senza risorse, che quindi non daranno questa ulteriore spinta, ed è un peccato. Aggiungo un altro elemento che mi sta particolarmente a cuore, perché so che il Ministero ha lavorato a un tavolo per l'istruzione e la formazione professionale,

L'istruzione e la formazione professionale affidate alle Regioni però non sono omogenee su tutto il territorio nazionale.

forse servivano risorse aggiuntive, per aiutare anche le Regioni a far partire più percorsi di istruzione e formazione professionale o quantomeno a creare quella programmazione creare quella programmazione che oggi non c'è. Voi qui parlate del quarto anno di istruzione e formazione professionale, ma sapete che, in tantissime Regioni, si è fermi ancora al terzo? E diventa difficile, poi, se non c'è un adatto ed adeguato finanziamento, arrivare tutti allo stesso livello. qui, una piccola chiosa: vanno messe in atto misure, che non si possono fare a costo zero, tali per cui i ragazzi che vanno in quegli istituti di istruzione e formazione professionali abbiano davvero la possibilità di completare in maniera serena il loro percorso. vero infatti che non tutti apprendiamo allo stesso modo, le fatiche sono tante e differenti. Questo percorso si propone di creare una scuola a misura di studente, ma, senza risorse, i ragazzi più fragili, come ricordava prima professor Crisanti, rischiano di rimetterci ancora di più, perché rischiano di non veder raggiunto l'obiettivo che sulla carta è scritto, ma che, senza alcun intervento aggiuntivo, rimane un'utopia il MoVimento 5 Stelle esprime, nel merito, un parere negativo su questo provvedimento, che tocca un tema assolutamente importante, come quello del raccordo tra istruzione e lavoro, ma in questo caso, lo fa, a nostro avviso in modo frettoloso, incompleto e superficiale. Il disegno di legge n. 924 tratta appunto il tema dell'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il ruolo della scuola e ponendolo in una funzionalità purtroppo subordinata. Diciamo subito che l'accelerazione impressa al provvedimento affinché possa partire già dall'anno scolastico 2024-2025 è un errore, che abbiamo provato a evitare presentando diversi emendamenti. Un nostro emendamento, tra i tanti che abbiamo presentato per provare a migliorare il testo,

approfondimenti il tema, presentato anche da altre forze politiche di minoranza, è stato bocciato, quando invece avrebbe dovuto indurre a una riflessione seria sull'evidente problema di tempistica rispetto alla possibilità di scelta che studentesse e studenti dovrebbero poter maturare. La fretta, signor Presidente, non è mai una buona consigliera e questo provvedimento arriva in Aula con troppa fretta. Il suo *iter* non gioverà certamente a trasformazioni di tale portata.

perché si va nella direzione sbagliata dell'impoverimento dell'impianto culturale del sistema di istruzione, sia perché l'obiettivo, in astratto condivisibile, di raccordare meglio l'istruzione con il mondo del lavoro viene attuato in questo testo con una metodologia affrettata, pericolosa e lacunosa. Molti percorsi scolastici risulteranno ridimensionati, come nel caso della riduzione sperimentale a quattro anni dei percorsi d'istruzione quinquennale. La domanda è: può essere questa una soluzione?

Presidente, per comprendere quanto nel nostro Paese ci sia bisogno di più scuola e non di meno scuola, basta ascoltare i ragionamenti di alcuni Ministri di questo Governo: basta ascoltare il ragionamento che fa il Ministro che parla di sostituzione etnica per capire che abbiamo bisogno di più scuola, non di meno scuola basta ascoltare lo stesso Ministro parlare del fatto che i poveri mangiano meglio dei ricchi per capire quanto abbiamo bisogno di scuola in questo Paese basterebbe il ragionamento che fa il Ministro della cultura, secondo il quale Dante Alighieri sarebbe il fondatore del pensiero della destra italiana: quest'affermazione, oltre a farci capire che abbiamo veramente bisogno di tantissima scuola in più,

più formazione con minor tempo a scuola, principio che chiaramente non potrà funzionare. Guardi, Presidente, non voglio nemmeno ipotizzare che questa devastazione della scuola italiana avvenga esclusivamente per creare manodopera a basso costo,

Con la frase «in funzione delle esigenze specifiche dei territori», questo provvedimento divide ancora di più il sistema scolastico italiano, che già subirà drammatiche conseguenze dallo scriteriato progetto dell'autonomia differenziata. Basti pensare che gli istituti tecnici superiori (ITS) sono situati prevalentemente nelle grandi Regioni, mentre nel Molise, in Umbria e in Basilicata c'è n'è soltanto uno. La scuola dovrebbe essere lo strumento migliore che il Paese ha a disposizione per garantire pari opportunità alle nuove generazioni e per ridurre le disuguaglianze generate dalle diverse realtà e opportunità territoriali. La scuola ha il ruolo di fornire ai giovani le competenze intellettuali e operative capaci di accompagnare le tante mutazioni che il mondo sociale e quello produttivo dovranno vivere. Per questo è fondamentale che mantenga sempre uno sguardo ampio e alto. Tale sperimentazione - perché è di questo che stiamo parlando - onestamente ci preoccupa non poco, perché pare voler anticipare un pericoloso percorso di riforma sostanziale dell'istruzione secondaria, nazionale e regionale, che avrà ripercussioni anche su quella terziaria, visto che ne modifica le forme di accesso, addirittura con la previsione di accesso agli ITS di studenti non solo con tipologie e livelli di formazione estremamente diversi, ma alcuni con l'esame di Stato superato e altri senza, con conseguenti diversificazioni negli eventuali percorsi successivi. Uno dei rischi è che percorsi così abbreviati e impoveriti producano l'effetto di una complessiva percezione di inutilità dello studio, di uno svilimento del tempo passato a scuola e della complessiva perdita di senso dell'istruzione in luogo di un precoce accesso al lavoro. La cultura del lavoro è uno strumento importante per fare scuola, ma viene svilita, se ridotta a singole esperienze proposte precocemente ad allievi che ancora non hanno sviluppato competenze di base e un'adeguata consapevolezza dei propri interessi e attitudini. Noi non siamo certamente contrari in assoluto al fatto che le scuole formino gli studenti anche rispetto a professioni specifiche, magari per un inserimento lavorativo più agevole, ma le modalità con le quali lo si sta facendo ci trovano in totale disaccordo, poiché sbrigative e controproducenti. Il modello proposto rischia di essere un *boomerang*, tra l'altro, anche per il mondo imprenditoriale, perché la spinta ad accompagnare precocemente gli studenti verso il mondo del lavoro, ben prima che acquisiscano i saperi e le conoscenze che rappresentano il presupposto di abilità e competenze specifiche, è contraria anche ad una politica di sviluppo che richiederà, in un mondo sempre più complesso e globalizzato, l'impiego di lavoratori più consapevoli e meglio formati. E che succederà, Presidente, se l'unica professione per la quale un nostro studente si sarà formato sarà tra quelle sostituite dall'intelligenza artificiale? Quale sarà il suo futuro, se avrà ricevuto una carente formazione scolastica? Al Al massimo, potrà fare il Ministro della cultura in questo Governo, ma non vedo tante altre alternative. *(Ilarità. Applausi)*. Quali sarebbero quindi i presunti benefici di questo provvedimento? Per la scuola pubblica, praticamente nessuno, mentre ci saranno per gli enti privati e per le imprese, in un disegno complessivo di privatizzazione dell'istruzione sempre più preoccupante. Noi ribadiamo con grande forza che si tratta di un processo che minaccia il sistema nazionale d'istruzione e che è doveroso fermare. Peraltro, per capire le sorti di questo progetto basta guardare i dati delle precedenti sperimentazioni

Si dimostra quindi chiaramente che le istituzioni scolastiche che hanno fatto esperienza diretta di un modello di scuola impoverito non lo hanno considerato efficace e di conseguenza lo hanno abbandonato. In conclusione, signor Presidente, secondo noi questo è un disegno di legge sul quale si doveva cercare una più ampia condivisione con il mondo della scuola, rimandandone nel frattempo l'attuazione. Invece, si sono di fatto respinte quasi tutte le proposte emendative sostanziali della minoranza in nome del principio del facciamolo subito e facciamolo male, che è ormai la consueta cifra stilistica di questo Governo. Per questo provvedimento ringrazieranno i privati, chiaramente a discapito del sistema scolastico pubblico, che è un po' quello che accade anche con la sanità. Il ministro Valditara disse mesi fa la seguente frase: «L'umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità». Vorremmo dire al Ministro dell'accorpamento delle scuole, al Ministro della perenne strizzata d'occhio ai privati, che è anche Ministro della scuola, purtroppo, che, se il suo obiettivo è quello di umiliare la scuola pubblica, purtroppo ci sta riuscendo alla grande. Signor Presidente, con questo provvedimento voluto dal ministro Valditara si interviene in modo concreto in una sfida strategica per il nostro Paese, per il suo tessuto produttivo e per il suo sistema formativo. Dobbiamo ammettere infatti che il nostro sistema formativo al momento non è sempre in grado di formare adeguatamente proprio le professionalità maggiormente richieste dal nostro sistema produttivo, che eccelle per caratteristiche di innovatività e intraprendenza note in tutto il mondo. Questa riforma, frutto anche del leale confronto con le Regioni, nel corso di un proficuo percorso legislativo in Commissione, costituisce una tappa fondamentale per la realizzazione di un progetto ambizioso e innovativo, rivolto a studenti e imprese, in grado di ridurre questo divario ereditato da un sistema formativo professionalizzante ormai obsoleto. L'istituzione della filiera tecnologico-professionale ha la finalità di ampliare l'offerta formativa a beneficio delle giovani generazioni attraverso un'integrazione tra il sistema formativo statale, principalmente consistente negli istituti tecnici e professionali, ma non solo, e quello della formazione professionale regionale, il tutto con il coinvolgimento fattivo del sistema delle imprese. Il cuore della riforma è rappresentato dalla costruzione di una filiera quattro che significa che i quattro anni di istruzione tecnico-professionale saranno collegati, anche dal punto di vista del percorso formativo, con il biennio degli ITS. Essendo il percorso di quattro anni, si potrà accedere prima agli ITS, ma anche all'università o direttamente al mondo del lavoro, senza che questo comporti una diminuzione della preparazione. La riforma punta, infatti, da una parte, al rafforzamento delle materie di base, come italiano, matematica e inglese, nelle quali oggi la formazione tecnico-professionale ottiene risultati sicuramente meno soddisfacenti rispetto alla formazione liceale e alle esperienze straniere,

ci saranno più docenti a disposizione degli studenti, potendosi così personalizzare la formazione sempre di più proprio nella direzione voluta dal Ministro, anche con l'introduzione del docente *tutor*. non si tratterà, come nelle precedenti sperimentazioni, di una semplice compressione dei programmi quinquennali in quattro anni, ma di programmi nuovi, pensati per le nuove esigenze didattiche e formative. si tratterà di una formazione di maggior qualità, in quanto più mirata, in grado di assicurare sbocchi professionali più qualificati in minor tempo. La stretta connessione con il sistema delle imprese passa poi attraverso due elementi: il ricorso all'apprendistato formativo di primo livello e il potenziamento del sistema alternanza scuola-lavoro e delle forme di inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studenti con disabilità. Il percorso sperimentale è particolarmente innovativo, perché darà più opportunità lavorative di maggior successo professionale ai nostri giovani, che troveranno più velocemente lavoro e al tempo stesso consentirà al mondo produttivo di essere più competitivo. Il disegno di legge contiene altresì un'importante passaggio, che consente di arricchire le specializzazioni laddove manchino i profili necessari tra i docenti. Le scuole potranno stipulare contratti diretti con imprenditori, tecnici o *manager* perché salgano in cattedra per insegnare ai ragazzi. Le novità poi riguardano le attività formative in lingua straniera, la promozione di accordi di partenariato, la valorizzazione delle opere dell'ingegno e il trasferimento tecnologico verso le imprese. Nella riforma, l'internazionalizzazione, infatti, giocherà un ruolo chiave, con collegamenti con istituti all'estero, *stage* e attività formative sulla base delle migliori esperienze europee. Le novità descritte troveranno immediata applicazione con riferimento ai percorsi quadriennali già avviati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo alla filiera formativa attivato per l'anno scolastico 2024-2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito. Ricordo infatti che questa riforma legislativa intende consolidare una sperimentazione avviata dal Ministro, in modo che questi percorsi possano essere attivi già dal prossimo anno scolastico. questa legge avrà certamente una sua effettiva e rapida attuazione: sono già 176 gli istituti tecnici e professionali che hanno avviato una sperimentazione che attende la consacrazione di questa riforma legislativa per dispiegare tutti i propri effetti. La concreta attuazione della filiera passa dal necessario coinvolgimento delle Regioni, a cui compete, come noto, la programmazione dell'offerta formativa sul territorio e il disegno di legge valorizza al massimo questo ruolo. Alle Regioni è rimessa la piena libertà di aderire e di definire in concreto le modalità realizzative, al fine di integrare e ampliare l'offerta formativa in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Per riorganizzare l'offerta formativa viene prevista anche la possibilità di costituire reti denominate *campus,* in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte. Per dare un segnale concreto e tangibile a supporto della realizzazione della filiera, si è prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni per il 2024 e cinque milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la progettazione degli interventi infrastrutturali. L'approvazione di un emendamento della Lega, infatti, segna un'innovazione anche di tipo infrastrutturale: i *campus*, dunque, quali luoghi di elezione per questa formazione integrata, potenzialmente aperti a tutti i gradi e le forme di istruzione collocati in quei distretti che si caratterizzano per la loro innovatività. Con questo fondo di complessivi 20 milioni si mette a disposizione delle realtà più intraprendenti del nostro territorio un patrimonio anche di risorse necessarie per la loro progettazione. Con questa riforma, dunque, si compie un passo avanti determinante per la modernizzazione del Paese, nella piena convinzione che il suo sviluppo debba passare dal rinnovamento dei suoi sistemi formativi, dall'ampliamento delle possibilità di scelta a beneficio dei nostri studenti e dalla piena sinergia con la parte più attiva e intraprendente del suo sistema produttivo. Di questo, come Gruppo Lega, ringraziamo sicuramente il ministro Valditara e personalmente ringrazio il presidente Marti e i colleghi della 7a Commissione, che non hanno fatto mai mancare il loro contributo all'esame di questo provvedimento. Signor Presidente, questo provvedimento del Governo avrà effetti molto pesanti e strutturali sulla nostra scuola e sulla nostra società, eppure ancora una volta è completamente calato dall'alto, senza condivisione con il mondo dell'istruzione, che subirà un impatto deformante con ripercussioni molto negative. Non è un caso che il Consiglio superiore della pubblica istruzione abbia espresso contrarietà; non è un caso che la gran parte degli organi collegiali delle scuole in ogni parte d'Italia (anche quelle a maggior trazione economica o manifatturiera), collegi dei docenti e consigli d'istituto, abbiano detto no alla richiesta pressante che viene dal Ministero per aderire immediatamente alla sperimentazione della riforma. Ci sono stati casi di forzature che hanno violato regole e statuti della democrazia scolastica e degli organi collegiali. In particolare, a dire no sono gli studenti, perché questa che voi, signori del Governo, chiamate riforma in realtà - ecco il rischio che vediamo - può scardinare un principio fondamentale del diritto allo studio, cioè l'eguaglianza nelle scelte e nell'accesso al sapere. Noi in Commissione cultura abbiamo dovuto insistere perché si tenessero almeno le audizioni su un provvedimento così impattante. Eppure, durante la discussione parlamentare, con uno sfregio evidente per gli auditi e per le scelte dei parlamentari, è arrivato il decreto del Ministro a silenziare, di fatto, tutti. Invece quelle audizioni sono voci fondamentali e vanno ascoltate, signor Presidente. Noi denunciamo il rischio che questo provvedimento scardini l'impostazione della scuola com'è scritta nella nostra Costituzione: una scuola per tutti, pubblica, universale e inclusiva. Questo atto rischia di spezzare in due il sistema dell'istruzione. Viene detto, con enfasi, con tutta la retorica della propaganda, che questa filiera formativa, tecnologica e professionale sarà innovativa. Noi pensiamo che non sarà così, intanto perché si tratta dell'ennesima riforma a costo zero: non c'è neanche un euro per i ragazzi o per i progetti didattici; gli unici fondi che vengono stanziati sono per una fantomatica struttura tecnica per la promozione della filiera. Ecco, ancora una volta, solo propaganda. Dite che gli istituti tecnici e professionali - che voi giudicate di serie B - domani diventeranno di serie A. Niente di tutto questo è vero, perché non c'è niente di innovativo nel ridurre il tempo scuola, nell'abbassare la qualità degli apprendimenti, nell'impoverire la preparazione complessiva degli studenti, nel rendere rigidi, senza alternative e già predeterminati i percorsi di sbocco per gli studenti, come ai tempi di quella che fu la scuola dell'avviamento prima del 1962. Qui c'è un "avviamento 2.0", altro che innovazione. Utilizzate parole altisonanti come «*campus*», ma in realtà c'è il rischio di cancellare conquiste sociali fondamentali. Si tratta di un modello regressivo che, di fatto, rischia di servire solo a fornire alle imprese manodopera a basso costo. È un modello che non contrasterà né dispersione scolastica, né povertà educativa. Per questo, la mia opposizione. Qui voglio esprimere un no forte e determinato e un no politico a questo provvedimento e a un'idea di Paese in cui a studiare e ad andare avanti sono solo coloro che già sono avanti, perché vengono da famiglie forti e benestanti, mentre la gran parte dei ragazzi, che vengono da famiglie che ogni giorno fanno i conti con le difficoltà, con la precarietà e con la crisi sociale, rischiano di non avere scelta di futuro e di non avere possibilità se non dentro un contesto che è già deciso da altri. Questo rischia di essere un ennesimo muro che impedirà a migliaia di ragazzi di accedere al sapere, che è un grande patrimonio sociale a cui tutti devono avere diritto, in particolare nel tempo che viviamo, quello di una piena e sconvolgente rivoluzione tecnologica. La scuola non è e non può essere una mera succursale del lavoro, di più se è un lavoro che rischia di essere dequalificato, precario e sottopagato. Con questa riforma viene introdotto di fatto un apprendistato senza retribuzione, i ragazzi devono sottostare, aumentando le ore di alternanza scuola-lavoro. Il rischio - lo voglio ribadire - è di avere manodopera formata, ma a basso costo. Presidente, dopo il colpo mortale dell'autonomia differenziata, anche qui viene prefigurata la fine del sistema di istruzione nazionale, disgregato in tanti circuiti locali, con differenze enormi da territorio a territorio. La scuola che viene qui definita non ha più un rapporto di primazia, di promozione nei confronti degli altri soggetti della società territoriale, com'era nelle intenzioni dell'autonomia scolastica. qui viene svuotata completamente quell'impostazione e viene imposto un modello subalterno, piegato completamente alle esigenze del mercato e delle imprese, con anche in cattedra esponenti di aziende, che non hanno i requisiti per insegnare. Attenzione, Presidente, nessuno di noi disconosce l'importanza del mercato e delle imprese, ma qui il tema è non svendere la scuola pubblica le sue potenzialità sociali e non barattare il destino di tanti ragazzi. Ridurre il numero di anni di studio metterà strutturalmente a rischio - checché se ne dica - organici e didattica. Ridurre il numero di anni di studio significa di fatto dequalificare, far calare il grado d'istruzione dei giovani. Questo acuisce diseguaglianze, disparità e discriminazioni sociali in un Paese - il nostro - in cui la scuola non è più un ascensore sociale e la parola merito, che voi avete messo a propaganda del vostro Ministero, in realtà significa privilegio. Non c'è niente di peggio infatti che dare di meno a chi ha già di meno, come qui si sta facendo. La disoccupazione giovanile in Italia oggi non è causata dal fatto che manchi una formazione funzionale alle imprese, ma dal fatto che spesso è impossibile trovare un'occupazione dignitosa e che l'offerta di lavoro è molto scarsa e perlopiù precaria e sottopagata. Noi diciamo che serve una scuola che sappia colmare il divario di partenza. Qui invece voi fate il contrario: acuite e rendete immodificabile Già oggi la gran parte delle scelte scolastiche dei ragazzi non dipende da inclinazioni, passioni, volontà, desideri singolo, ma dalla collocazione sociale dei genitori. I figli di alcune famiglie vanno al liceo. I figli della gran parte delle altre famiglie vanno negli istituti tecnici e professionali. Nella gran parte dei casi non è una scelta libera, ma condizionata. I primi poi andranno all'università e ambiranno ad alcuni ruoli sociali. I secondi, tendenzialmente, non potranno andare all'università, come rilevano già ora le statistiche, e si vedranno precluse possibilità e opportunità. Questa che chiamate riforma certifica una barriera di censo e di classe, spaccia per modernità e innovazione qualcosa di molto vecchio, che abbiamo già conosciuto. È un passo nel passato, che pregiudica diritti fondamentali, conquistati in anni importanti della nostra Repubblica. Per questo, Presidente, dico qui il mio no.

al ministro Valditara, alla relatrice Bucalo e chiaramente anche al presidente della 7a Commissione Marti, che ha consentito che questo provvedimento

veramente una strada nuova per gli studenti. Apre una strada nuova, dopo tanti anni che si dice che la scuola rimane solo una formazione fine a sé stessa e che non prepara gli studenti al mondo del lavoro. Nel momento in cui arriviamo a deliberare un provvedimento in questo senso, chissà perché nascono mille problemi, mille paure e mille contraddizioni, oserei dire. Finalmente invece oggi diamo una strada e apriamo un'opportunità, attraverso questo corso quadriennale, per far sì che gli studenti arrivino già preparati in un certo mondo del lavoro,

si è voluta creare una condivisione con l'impresa e con il mondo del lavoro, un qualche cosa che fino adesso non avveniva. In questo senso il Governo sta dimostrando attenzione concreta nella formazione degli studenti al mondo del lavoro (si veda anche il liceo del *made in Italy*). Ebbene, prendo alcuni spunti che i colleghi intervenendo mi hanno dato, nel criticare l'istituzione della filiera tecnologico-professionale. Parto da ultimo con il senatore Verducci, quando parla di manodopera a basso costo. Non so in base a quali principi asserisca questo, faccio fatica francamente, con tutta la buona volontà, a capire cosa c'entri la manodopera a basso costo con l'istituzione della filiera tecnologico-professionale. fine coerentemente dice: «Il mio è un no politico». Allora, nel rispetto ideologico accettiamo anche il no politico; diverso è invece il no nel merito di questo provvedimento.

ai privati; si dice che è una scatola vuota, si dice che è supportato dalle *lobby*, si dice che è un marchio di disuguaglianza, si dice che è di proporzioni allarmanti.

Si parla poi di disomogeneità sul territorio di questa formazione, in quanto, per ovvie ragioni, ogni Regione ha una sua storia e ogni Regione ha un suo tessuto industriale che la caratterizza, ma non la sminuisce rispetto ad altre aree del territorio nazionale. Anzi, se volessimo vederla in senso positivo, anche nella logica dell'autonomia differenziata che abbiamo

per il proprio territorio. Questo non è negativo, ma è assolutamente positivo. Cito altri colleghi, per dire che questa non omogeneità, casomai ci fosse, è un valore aggiunto.

formativi, innovativi verso la formazione dello studente, focalizzato poi ad inserirsi nel mondo del lavoro. Prendo infine ad esempio quanto detto dalla senatrice Malpezzi.

apre una nuova finestra"). Dichiaro chiusa la discussione generale. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.

perdita per le istituzioni scolastiche del ruolo di titolarità rispetto al rapporto con le aziende e le realtà produttive del territorio, che non vi è nessuna possibilità di scelta per i ragazzi. Ebbene, signor Presidente, questi non sono problemi, anzi, direi che sono problemi legati solo ad un retaggio culturale sbagliato. tempi di approvazione, nel mese di gennaio del 2024 si è raggiunta la quota del 49 per cento tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro, mancano figure specializzate nel campo dell'industria tessile e delle confezioni. Siamo arrivati ad una percentuale del 72 per cento di figure specializzate ricordo a me stessa e ai colleghi che il nostro è il secondo Paese in Europa nel campo della manifattura.

Stiamo parlando di settori importantissimi di traino per la nostra economia che sono indietro sia nella produzione, sia nella consegna, con un mancato PIL pari a 38 miliardi di euro. Di contro, ci ritroviamo con un tasso di disoccupazione giovanile del 20 per cento, quindi di cosa stiamo parlando? di cosa stiamo parlando? Questo è un provvedimento necessario, è un provvedimento che ha avuto la forza e la capacità di cogliere al volo il grido delle nostre imprese, del nostro mondo produttivo. i ragazzi non hanno nessuna possibilità, ma aver coordinato la sperimentazione e il un vantaggio per loro, perché già per il prossimo anno scolastico possiamo dire che questa legge avrà una più rapida attuazione. In 171 istituti tecnici e professionali, sono stati avviati corsi in sperimentazione che si caratterizzano soprattutto per le progettualità innovative e per il concreto coinvolgimento del territorio e delle imprese. E voi mi dite che questo non è un beneficio per i nostri ragazzi? Ma è evidente che tutto questo è il futuro per i ragazzi, è una possibilità importante per il loro futuro. data dal carattere quadriennale della sperimentazione. Sappiamo tutti che i nostri giovani arrivano nel mondo

purtroppo, ha il primato negativo nell'Unione europea per giovani inattivi. Cosa si è fatto in tutti questi anni se non offrire strumenti basati sull'assistenzialismo, dando ai nostri ragazzi solo il reddito di cittadinanza? Non c'è stata una possibilità intelligente di formarli, capace di dare ulteriori possibilità di un futuro lavorativo, di avere in tempi brevi ragazzi ben formati e soprattutto capaci di trovare un posto di lavoro. *(Applausi)*.

n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

il parere è favorevole a condizione che si sopprimano le parole: «e alla cultura generale».

si prende tutto il tempo necessario per trovare un accordo, che non hanno anche su un provvedimento semplice. *(Applausi)*. Dopodiché, sempre sull'ordine dei lavori, dato che questa è sempre l'Aula del Senato, il Governo, la maggioranza e la relatrice danno un parere, quello è il parere. Non è che il parere si cambia. Noi abbiamo aspettato i due minuti e abbiamo ascoltato anche il cambio di parere. Ci augureremmo che d'ora in poi la relatrice ci fornisse dei pareri stabili, anche perché sono corroborati dal parere del Governo. Immagino che anche la sottosegretaria Frassinetti stia cambiando i pareri. Questo non mi consola, perché vuol dire che non c'è una grande certezza.

nazionali. Io non riesco a capire perché tutti gli altri ordini di scuola devono avere linee guida nazionali e, rispetto a questo progetto, non lo dobbiamo ribadire. O mi si dice che è pleonastico, ma me lo si conferma in qualche modo; altrimenti qualche dubbio a me viene. Siccome non costa, mi dovete spiegare perché gli altri indirizzi avranno linee guida nazionali e questi no.

stabilite dal Ministero dell'istruzione e del merito. Anche in questo caso, perché non deve esserci il rispetto delle linee stabilite dal ministro Valditara? In questo momento è lui chiamato a stendere queste linee. Io vorrei capire per quale motivo non siete d'accordo su questo punto. Nel rispetto dell'autonomia, poiché nessuno vieta alle filiere di avere la propria natura legata al territorio, su dei punti chiave, però, la formazione dovrebbe essere comune da Nord a Sud, nel rispetto delle curvature delle singole scuole. Per quale motivo non c'è una base nazionale comune scritta dal Ministero dell'Istruzione del merito? Il ministro Valditara è assente oggi. Ci sarebbe piaciuto fare a lui questa domanda, ma evidentemente non vuol venire

e vorrei che fosse spiegata. Questo emendamento dice una cosa semplicissima: il provvedimento consente alle filiere di stipulare dei contratti esterni con figure professionali di altri mondi, che può essere una cosa anche utile: se hai bisogno dell'esperto in un determinato settore, va bene. Dopodiché, però, l'emendamento a prima firma Camusso dice una cosa logica, che si sposa con tutto ciò che è già scritto nel testo. Nel testo ci è stato detto - e di questo siamo contenti e avremmo voluto che fosse esplicitato maggiormente che comunque non ci sarà un calo nell'organico, perché dai cinque anni i percorsi scendono a quattro, ma saranno rimodulati e non ci sarà né esubero di personale, né diminuzione dell'organico nelle scuole. Questo è scritto nel testo.

questa maggioranza che, rispetto alle graduatorie, ha una posizione quanto mai schizofrenica. Tutte le volte che dicevamo che ci voleva il concorso e che le graduatorie dovevano essere esaurite,

che, quando hanno potuto, hanno assunto, hanno dato stabilità al personale della scuola e hanno cercato di ridurre le graduatorie con il più grande piano di assunzione. E ce lo dovremmo ricordare tutti. Qui addirittura si dice che, nonostante ci possano essere degli spazi, quelle graduatorie non devono essere considerate. Penso sia un grosso errore o una grossa ambiguità.

nell'ultima pagina del fascicolo degli emendamenti in distribuzione.

Vi leggo il parere sul testo e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche all'articolo 4, sopprimere le parole: "delle proiezioni"; sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026"; sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".

mettendoci zero euro. Gli unici soldi che ha messo, quelli per cui poco fa abbiamo visto la rimodulazione annuale, nascono da un emendamento del presidente della 7a Commissione Marti per la costituzione dei *campus*. Ma a favore degli studenti, dell'offerta formativa e dello sviluppo anche della formazione professionale, che

professionale, noi oggi avremmo fatto un lavoro migliore per la scuola. Come ribadisco, questo provvedimento a disposizione delle scuole e quindi dell'offerta per i ragazzi non mette un centesimo.

Grazie,

tecnico secondaria presentata dal ministro Valditara, la cosiddetta 4+2, è l'ultimo tassello di un *puzzle* più ampio che riguarda la filiera della formazione tecnica e delle scienze applicate del nostro Paese; una filiera costruita su tre pilastri che sono - lo ricordo - la riforma degli ITS - è stata approvata all'unanimità nella scorsa legislatura, e aveva, tra i primi firmatari, l'ex parlamentare Serse Soverini - la riforma dell'orientamento scolastico e la 4+2. La valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale serve ad assicurare competitività al Paese qualità ai nostri giovani, superando uno stigma radicato nel nostro Paese che scoraggia gli studenti a scegliere i percorsi dell'istruzione tecnica. Vorrei che su questo chi ha responsabilità politiche si assumesse la responsabilità, perché per anni noi abbiamo considerato quella tecnica un'istruzione di serie B. Questi provvedimenti servono invece a restituire dignità e qualità agli insegnanti e agli studenti che partecipano ai corsi di istruzione tecnica. Quando la legge sugli ITS, che ricordo era stata voluta dal Governo Draghi e rientrava nelle riforme previste dal PNRR per avvicinare il nostro sistema a quello duale, a quello tedesco, in Assemblea si era raggiunta l'unanimità. Ecco, io mi chiedo, per coerenza con quel percorso che vede nel 4+2 un tassello di questa riforma, non avremmo avuto forse più coraggio se avessimo accolto le proposte che oggi ci vengono fatte dal ministro Valditara o solo perché vengono fatte da questo Governo o dal ministro Valditara non dovrebbero essere accettate?

che, in questo caso, si chiama il diritto alle competenze dei giovani, che noi crediamo debba essere riconosciuto come diritto fondamentale delle persone. Noi parliamo di transizione digitale e di transizione ecologica. Sappiamo quante risorse il PNRR prevede per la transizione ecologica e per la transizione digitale.

che il tema dell'istruzione si avvicini ai temi richiesti dal mercato del lavoro? Voi sapete che l'85 per cento dei ragazzi che esce da questi percorsi trova uno sbocco professionale. Ho sentito parlare di svendita dell'istruzione ai privati e alle imprese. Noi rinneghiamo questa visione ideologica riteniamo che invece si stia lavorando per affermare la qualità dell'istruzione tecnologico-professionale per affermare il diritto alla competenza dei nostri giovani. Abbiamo presentato degli emendamenti e ringrazio

sono deceduti perché il problema della sicurezza in Italia riguarda il lavoro, i luoghi dove il lavoro si svolge, ma riguarda anche quei laboratori in cui si svolgono i tirocini, gli *stage* e i percorsi curriculari. abbiamo chiesto di potenziare il tema linguistico, il tema delle competenze matematiche e - perché no? - il tema della cultura generale. Ci dovrete poi dire perché la cultura generale no e l'altra competenza linguistica matematica sì. Accettiamo però l'apertura che c'è stata fatta. un terzo tema affrontato dagli ordini del giorno, uno a firma della collega Versace che parla dell'accessibilità dei laboratori. Voi sapete quanti di questi laboratori siano inaccessibili. riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Io mi chiedo: ma se stiamo parlando di una riforma sperimentale, se stiamo parlando di corsi sperimentali, come possiamo non immaginare dei corsi che prevedano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per gli studenti e per gli insegnanti, laddove questo non è il futuro, ma è già il presente della nostra formazione?

sperimentali quadriennali della filiera tecnico-professionale. Arrivo alla conclusione, Presidente. Azione voterà a favore di questo disegno perché, coerentemente con l'impegno già assunto in precedenza, noi siamo a favore del diritto alle competenze dei giovani, siamo per creare le competenze che ci servono per avere qualità nell'istruzione secondaria e siamo anche per sostenere un percorso di riforma dell'istruzione tecnica secondaria, che oggi con il 4+2, dopo l'ITS e dopo l'orientamento, arriva a compimento.

In un Paese peraltro come il nostro, dove non sono ancora sufficienti gli investimenti per innalzare i livelli di istruzione, il Governo, piuttosto che provare a contrastare grandi e annosi problemi come la dispersione scolastica e le non raggiunte competenze di tanti di fronte al dilagante disagio giovanile, che si concentra soprattutto nelle periferie, ci propone un modello di scuola che vorremmo definire di "scuola meno".

visto che gli esiti di tutte le esperienze precedenti che sono state avviate hanno mostrato uno scarso consenso verso i percorsi quadriennali, sia tra gli studenti sia tra i genitori, ma anche nelle stesse istituzioni scolastiche a cui sono state poi effettivamente indirizzate le sperimentazioni. dai dati ministeriali che soltanto 243 scuole sulle 1.000 che erano state previste hanno chiesto di sperimentare il modello del diploma in quattro anni e che le 192 sperimentazioni avviate a seguito del decreto-legge n. 89 del 2 febbraio 2018 sono passate a 175 classi già nell'anno scolastico successivo e ad oggi i rinnovi si sono ancora ridotti e sono diventati 98. Insomma, si dimostra chiaramente si dimostra chiaramente come le istituzioni scolastiche, che hanno fatto per l'appunto l'esperienza diretta di un modello di scuola ridotto, non lo hanno considerato efficace e di conseguenza lo hanno abbandonato. Sottolineo anche anche che sarebbe stato invece assai utile mantenere gli attuali percorsi quinquennali, soprattutto al fine di non impoverire l'offerta formativa rivolta a un settore costantemente sottoposto alla trasformazione delle tecnologie e alla frequente modifica delle operatività necessarie alla tenuta e allo sviluppo industriale ed economico. Le competenze acquisite diventano sempre più facilmente e rapidamente obsolete, come sappiamo, e pertanto appare, dal nostro punto di vista, assolutamente necessario curare in maniera molto approfondita il tema grande dell'acquisizione dei saperi e delle conoscenze che lo sostengono, in modo da poter contare in futuro su lavoratori e lavoratrici capaci effettivamente di confrontarsi con la complessità di tecnologie in costante trasformazione. Sarebbe stato quindi auspicabile cercare di rafforzare le esperienze laboratoriali che potessero anche valorizzare alcune specificità professionali, senza confondere però quello che la scuola ha il compito di fare, cioè educare e istruire e non invece ammaestrare

Presidente, aggiungo che non siamo certo noi gli unici ad essere in disaccordo con questa sperimentazione, perché le stesse organizzazioni sindacali e molte associazioni di categoria hanno espresso un forte disappunto. Anche nella fase della mia vita in

vorrei aggiungere un'ulteriore riflessione. L'assenza dei licei nel progetto sperimentale suggerisce, dal nostro punto di vista, una visione davvero totalmente classista della divisione tra l'istruzione liceale e quella tecnico-professionale, limitando i trasferimenti da indirizzi e percorsi, nonostante l'invocazione del concetto di *campus*. una questione, quella del classismo, sulla quale spesso ho richiamato quest'Assemblea a un elemento di attenzione, perché penso essere uno dei grandi temi che attraversano oggi la scuola italiana. Tante volte ho segnalato in quest'Aula come le statistiche con le quali abbiamo a che fare ci segnalino un problema gigantesco, cioè che la stragrande maggioranza degli studenti che oggi sono iscritti ai licei classici e ai licei scientifici provengono da famiglie nelle quali i genitori, a loro volta, sono diplomati ai licei classici e ai licei scientifici e accade esattamente l'opposto per gli istituti tecnico-professionali. Questo rappresenta un problema enorme, perché introduce un'idea che è esattamente il contrario di quell'ascensore sociale attorno al quale si era costruita e creata la nostra democrazia per molti decenni. Inoltre, alla luce dell'autonomia differenziata, l'inclusione dei percorsi delle istituzioni formative regionali richiederebbe anch'essa un'analisi approfondita, considerando più attentamente gli aspetti giuridici e normativi. Attualmente, chi completa il diploma professionale del quarto anno deve affrontare un anno aggiuntivo e deve sostenere l'esame di Stato per accedere agli ITS, che sarebbero gli istituti tecnici superiori. È evidente, almeno dal nostro punto di vista, che i percorsi della formazione professionale quadriennale attuale non sono equiparabili all'offerta formativa dell'istruzione tecnica e professionale, compromettendo l'efficacia complessiva della formazione. Anche in questo senso sarebbe davvero opportuno avviare la sperimentazione con un campione magari più limitato e prevedere l'istituzione di un vero e proprio monitoraggio.

con docenti stabili, che possano accompagnare gli studenti per tutto il percorso di istruzione, evitando il balletto degli insegnanti cui assistiamo ogni anno e che spesso colpisce gli studenti più fragili, in particolare i ragazzi disabili. Io non credo che ci sia bisogno di questa ennesima sperimentazione, che rischia di creare soltanto una inutile e dannosa sovrapposizione di percorsi. Per questo motivo esprimiamo un voto negativo, perché davvero pensiamo che investire sulla scuola, sull'istruzione e sulla formazione significhi investire sul futuro. E non mi stancherò di dire in quest'Aula che non l'abbiamo fatto sufficientemente nel corso degli anni passati, ma rischiamo, ancora una volta, di perdere una clamorosa occasione e di continuare a non farlo.

(se non felice, perché c'è troppo dolore nel mondo e nei nostri condomini per essere felici: non ce lo possiamo permettere, se non forse nell'intimità della nostra vita affettiva). Questo provvedimento era fortemente sentito, anzi, se potessi usare un neologismo, fortissimamente sentito, perché nessuno vieta, a chi si occupa di docimologia, di pedagogia, di industria e di investimenti nella salute culturale dei figli, anche con i propri sforzi nella vita quotidiana, di pensare ad un provvedimento che tenti, con tanta buona volontà, ma considerando un pregresso veramente complesso, di collegare

È uno strumento di percezione della realtà che da tanti anni si sentiva come necessità. Quante volte si è detto che negli altri Paesi si studia di meno, ma ci si collega di più con la realtà?

direttori d'istituto, degli insegnanti, del collegio dei genitori e della buona volontà dei ragazzi e delle ragazze,

queste due realtà nel terribile *post-*Covid (Covid gestito così male nel nostro pianeta Italia), c'è necessità più che di cambiare, di innovare la motivazione delle ragazze e dei ragazzi, degli insegnanti, ma anche di quello che sta fuori, dall'industria alla famiglia. famiglia. Nel provvedimento, tra l'altro, si prevedono convenzioni e collegamenti reali con le realtà regionali, mai vissute come antagoniste, antagoniste, Presidente, come credo che sia anche nell'autonomia differenziata, che anzi dovrebbe migliorare questa realtà. Io credo

dica sempre no. Io sono un affezionato dell'opposizione, l'ho fatta per anni, dal Comune alla realtà nazionale, e so bisogna anche fare le pulci a quello che viene considerato l'avversario vincente (avversario, ma non nemico). Se c'è un provvedimento come questo, che tra l'altro ha ascoltato le voci dell'opposizione, dico che, piuttosto che opporsi, occorrerebbe cercare di far applicare le norme nella realtà socioculturale del Paese, territorio per territorio, come qualcosa che tende a migliorare. Lo dico con esperienza antica (e forse qualcuno dirà che è talmente antica che è meglio che io smetta; forse è vero, ma finché non me lo dice la mia coscienza

quello che conta è anche non essere contro pregiudizialmente, ma cercare di impostare nella concretezza della quotidianità il provvedimento stesso Ho molta speranza che gli amministratori locali, chi gestisce gli istituti di formazione, i genitori e soprattutto le studentesse e gli studenti

frequento molto la scuola, che a me è stata negata, in quanto dicevano che avrei messo paura agli altri studenti, quindi ho dovuto trascorrere - tranne il liceo meraviglioso tutta la mia vita scolastica a casa e so cosa vuol dire l'emarginazione dalla cultura scolastica, dall'apprendimento e anche

banchi dedicati a chi sul momento gestisce un provvedimento, e mi sento un po' un ingombro.

quando sento parlare di persone con disabilità, fra cui me, mettendole in relazione al termine "fragili", con tutti il rispetto per chi lo pronuncia, una parte di me si ribella. La mia ribellione è molto pacifica, ma non per questo meno virulenta in me stesso. Noi non siamo fragili. Certo, siamo più esposti di altri a problemi legati a malattie, all'epidemiologia, possibilità di ammalarsi o di avere più difficoltà nel superare le barriere architettoniche, culturali e sensoriali, ma non siamo fragili. Noi siamo forti, perché sfido chiunque di voi ad affrontare - lo dico senza pietismi - la vita quotidiana con qualche disabilità vera e arrivare alla sera con serenità a gestire le persone che amano e dalle quali sono amate. Il diritto all'amore forse il diritto più negato, ma più forte, per il mondo della disabilità, con le sue mille configurazioni. Parliamo di persone con criticità, con difficoltà

una discussione ampia e un confronto completo su questo provvedimento. L'ottimo lavoro della relatrice, la senatrice Bucalo, ha consentito di ottimizzare tutti i contributi offerti dai senatori, inclusi quelli di opposizione. Il risultato è un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro e ai ragazzi che intendano seguire i percorsi formativi tecnologico-professionali. Si tratta di un testo fondamentale per migliorare la filiera professionale e tecnica, che da oggi viene messa sullo stesso livello di altri percorsi formativi. Peraltro, questo nuovo percorso avvia la sua fase sperimentale, cui seguiranno la verifica e il monitoraggio dei risultati. Questo è un provvedimento importante, che affronta il problema di far acquisire ai giovani le competenze concrete che richiede oggi il mondo del lavoro, quindi diventa fondamentale la promozione della filiera formativa tecnico-professionale. È importante anche investire nelle strutture e nei laboratori avanzati e innovativi per completare la didattica per gli studenti e per la loro formazione. Viene in questo modo valorizzato il valore formativo che può essere dato dalle Regioni, che hanno competenze precise sul tema, loro garantite dalla Costituzione. Con queste disposizioni, quindi, i percorsi di formazione professionale hanno un ruolo paritetico rispetto ad altri percorsi di istruzione secondaria. Per ora - è vero - si tratta di sperimentazione che avviene all'interno delle previsioni e delle tempistiche del PNRR, ma a questa sperimentazione può seguire un percorso di studi permanente, che vada in modo serio incontro alle esigenze del mondo delle imprese e che riesca a dare uno sbocco lavorativo immediato agli studenti che frequentano questo indirizzo scolastico. Con il provvedimento in esame investiamo sui giovani, investiamo sul futuro. Forza Italia, proprio per la concretezza delle norme di questo testo e dei percorsi di studio in esso delineati, che avvicinano la scuola e il mondo del lavoro, valuta positivamente questo disegno di legge e voterà in modo convinto a favore.

Quello che ci domandiamo, infatti, è se fate finta di non capire dove state portando i nostri giovani e il nostro Paese o se davvero vi manca totalmente la visione e quindi andate a mettere toppe peggiori dei buchi dove vi sembra che ci sia una necessità di intervento. Mi spiego meglio, cercando di argomentare. Perché dovremmo cambiare il numero di anni necessari ai nostri giovani per istruirsi e poi formarsi?

fare e c'è un periodo della vita in cui i nostri giovani li dobbiamo istruire; poi, chi non vuole proseguire, pensando di non avere bisogno di ulteriore istruzione, e preferisce indirizzarsi direttamente al mondo del lavoro, segue un percorso di formazione. Nel provvedimento in esame, invece, vedo che si cerca di ibridare i due percorsi e di solito queste cose non portano mai a nulla di buono. Forse volevate copiare il sistema duale tedesco, ma - come al solito male: neanche quando potete prendere ad esempio qualcosa che funziona, riuscite a farlo nella maniera corretta. Anche in quel caso, infatti, dopo il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria - i giovani possono essere indirizzati a un percorso di formazione e pratica, ma lo fanno avendo alle spalle un contratto di tirocinio lavorativo che prevede anche una retribuzione. Non so se avete una certa familiarità con questo termine, perché in qualche modo anche nel percorso di apprendistato il lavoro va retribuito

che male ci sarebbe? Pensate che ai genitori italiani dia fastidio mantenere i propri figli un anno in più e che ci sia tutta questa smania di mandarli a lavorare? Lo capisco, in un certo senso: avete tolto pure il reddito di cittadinanza a diciott'anni, quando l'istruzione superiore finisce a diciannove, quindi è chiaro che in ogni modo dovete cercare di sgravare le famiglie, secondo voi. Le famiglie non sono più quelle fragili, perché i figli devono andare a lavorare anni; l'ascensore sociale lo lasciamo agli altri, perché chi è povero deve continuare a fare il povero, magari pure sfruttando i figli dei poveri, mentre invece i vostri figli li mandiamo al liceo, magari privato, poi a fare un corso universitario, poi a fare il *master* all'estero. I vostri figli, infatti, sì che si devono istruire correttamente, i figli delle classi inferiori li mandiamo a fare l'istituto tecnico, gli accorciamo un anno e li spediamo subito, magari anche con un calcio nel didietro, a lavorare. *(Applausi)*. Questa è la visione di Paese che avete?

provvedimento arriva soprattutto dalle richieste del Nord-Est, dove le fabbriche sono affamate di manodopera da pagare sempre meno, perché, se si specializza di più, poi la dobbiamo pagare troppo. Soprattutto, mandiamo a lavorare i nostri giovani il prima possibile: non sia mai che poi ci serva manodopera e debba arrivare dall'estero; guai ad aver bisogno di manodopera dall'estero, vero? Dobbiamo Dobbiamo preservare la nostra etnia, ovviamente, perché il disegno poi si riconduce sempre agli stessi punti. Per non parlare poi anche dell'ossessione che avete nei confronti dei giovani che stanno sul divano per colpa del reddito di cittadinanza. Noi li vogliamo mandare a scuola e voi invece li volete mandare a lavorare. Guai a farli formare un po' meglio e guai ad avere un po' di istruzione: è ovvio che, se poi i giovani li istruiamo meglio, magari viene loro voglia di viaggiare, di visitare i musei, di acculturarsi, di staccarsi dalla televisione e da quei programmi, magari Mediaset, da pane e e donne un po' svestite con cui li volete crescere. Fate loro credere che a diciott'anni la cosa più bella sia andare a lavorare, guadagnare magari 1.000 euro, mentre ci mantengono i nostri genitori, avere la macchina per andare il sabato sera in discoteca; però poi non gli diciamo che quando avranno trent'anni continueranno a guadagnare 1.000 euro, perché non si sono formati abbastanza e da casa di mamma e papà non se ne potranno andare, perché con 1.000 euro una casa propria, un affitto e un futuro non se li possono costruire.

a volte si perde anche il filo del discorso, se si viene continuamente interrotti. *(Applausi)*. Quello che vorrei chiedervi è perché, invece di guardare al fatto che i nostri giovani vanno a lavorare più tardi, non guardate alle statistiche, che dicono che che i livelli di istruzione nel nostro Paese sono più bassi rispetto all'estero e che abbiamo meno laureati? È questo che vi dovrebbe preoccupare e non di averne ancora di meno, né tantomeno di creare discriminazioni tra gli studenti che frequentano un percorso scolastico rispetto ad un altro. Nel provvedimento infatti avete scritto che uno studente che fa questo percorso si può anche iscrivere all'università un anno prima rispetto al coetaneo che decide di fare un percorso lineare perché ha le idee chiare fin da subito sul fatto che voglia andare all'università.

che non appartengono al vostro vocabolario. Qualsiasi sia l'argomento di cui stiamo discutendo. Per non parlare poi di un altro vostro pallino, per non dire fissazione. Siccome non ci piacciono gli insegnanti che arrivano dal Sud ad insegnare nelle scuole del Nord, aprite anche ai contratti di prestazione ad opera per l'attività di insegnamento, senza concorso dal momento che questi contratti si fanno senza e sicuramente assumendo qualcuno che ci fa comodo e che sta vicino a noi nella nostra zona, con una residenza squisitamente nordica. Ovvio, ma certo, andiamo avanti così. Chissà cosa ne penseranno i sindacati della scuola e tutti gli insegnanti? Giusto per continuare a sottolineare che voi se visione avete, ce l'avete davvero localistica, individualista e classista. Questi sono gli aggettivi che vanno bene per voi. Ancora un altro provvedimento che blocca l'ascensore sociale nel nostro Paese, che impedisce la crescita crescita e il miglioramento collettivo. E voi sareste quelli che vogliono aumentare il PIL del Paese, lasciando fare a chi vuole fare? Secondo me non sapete dove ci state portando. *(Applausi)*. A sbattere sicuramente. Per tali ragioni il voto del MoVimento 5 Stelle sarà convintamente contrario. Presidente, ci apprestiamo a votare un disegno di legge di iniziativa del ministro Valditara, su cui nella Commissione che mi onoro di presiedere abbiamo lavorato con grande celerità, ma in modo altrettanto approfondito, certi che si trattasse di uno strumento necessario a valorizzare gli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica e professionale,

che si trattasse di uno strumento necessario a valorizzare gli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica e professionale, rendendoli più efficaci per sviluppare le competenze necessarie all'ingresso nel mondo del lavoro. Oggi si istituisce la filiera formativa tecnologico professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal PNRR, per potenziare l'offerta di servizi di istruzione in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche incentrate sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori. così finalmente una risposta alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0, la strategia di politica industriale del Governo per promuovere la digitalizzazione e il rafforzamento competitivo del tessuto produttivo italiano. Il Paese ha bisogno di misure tese a creare un ambiente attrattivo per gli investimenti anche all'estero e a incentivare la creazione e lo sviluppo di imprese ad alto valore tecnologico. Questa riforma costituisce un passaggio nevralgico e una leva importantissima per la crescita economica dell'Italia. I nostri ragazzi in quattro anni potranno ottenere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma agli studenti è assicurato il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Potranno poi proseguire con il biennio formativo presso l'ITS Academy per conseguire un titolo di alta specializzazione tecnica. È il modello 4+2, che rafforza il rapporto tra scuola e azienda, permettendo da un lato ai nostri ragazzi una formazione qualificata, che consentirà di accedere più facilmente al mondo del lavoro, e dall'altro alle imprese di avere professionalità altamente profilate e competenti. Sono orgoglioso, a nome anche del mio Gruppo, di aver contribuito con un emendamento al finanziamento di 15 milioni per il 2024 e di ulteriori 5 milioni per il 2025 e per il 2026 (quindi un importo totale di 25 milioni), per avviare la progettazione di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di veri e propri *campus* multiregionali e multisettoriali per favorire la formazione integrata, che è una delle principali finalità sottese da questo disegno di legge. Infatti dei *campus* possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e di formazione professionale (percorsi di IFTS e ITS Academy), le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli altri soggetti pubblici e privati, ivi comprese le imprese. *(Applausi)*. Si crea così l'opportunità di utilizzare alcune aree strategiche del nostro territorio nazionale, sviluppandone le potenzialità; aree che consentiranno di creare sinergie culturali e strutturali tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale, scientifico e tecnologico. Ma non dimentichiamo che i ragazzi potranno anche scegliere di iscriversi a qualsiasi corso di laurea. Finalmente avremo dei percorsi scolastici efficienti per sviluppare le competenze chiave necessarie per la vita e per l'ingresso nel mondo del lavoro, connessi con il mondo del lavoro e con un'attenzione particolare ai nuovi lavori e alle professionalità emergenti, attrattivi poiché basati su esperienze pratiche e laboratoriali, grazie all'apporto di lezioni e di attività laboratoriali tenute da esperti provenienti dalle aziende e dal mondo stesso del lavoro, aperti soprattutto alle opportunità di studio e di lavoro anche all'estero, con il rafforzamento delle competenze STEM e linguistiche. Questa riforma non impoverisce il sistema scolastico, come qualcuno dell'opposizione vuole paventare. Al contrario, questo provvedimento e questa riforma porta un arricchimento, perché forse c'è qualcuno che non ha letto bene questo testo, oltre anche a puntare sul rafforzamento delle attività laboratoriali e dell'alternanza scuola-lavoro. La riforma prevede a chiare lettere il rafforzamento delle competenze nelle discipline base, ovvero l'italiano e la matematica. Avremo lezioni personalizzate e *tutor*; così la formazione, la peculiarità e le esigenze di ciascuno studente potranno essere valorizzate a pieno. Sono anni e anni che la politica non dà risposte in questo senso. Il nostro Paese è in fondo alle classifiche europee per i giovani impiegati e per il *mismatch* fra domanda e offerta di lavoro. Ma con questo Governo abbiamo finalmente cambiato la rotta. È per questo che sono già tanti gli istituti che hanno aderito alla primissima sperimentazione, con il prossimo anno scolastico, e sono tantissime le iscrizioni raccolte, prima ancora della scadenza dei termini.

il disegno di legge che siamo chiamati a votare, la filiera tecnico-professionale, coinvolgendo i tecnici professionali, diversi percorsi di istruzione e formazione regionale e l'istruzione tecnologica superiore, avrà un impatto decisivo sul nostro sistema di istruzione. È dunque una discussione importante quella che stiamo facendo ed è un voto importante quello che siamo chiamati a dare, che noi non daremo in modo superficiale. Un voto importante su un percorso che avrebbe meritato, per un'efficace sperimentazione, un ripensamento dell'intero sistema, dei suoi *curricula* e delle modalità didattiche, pena il rischio di un salto nel vuoto, con un indebolimento complessivo del livello di formazione delle nuove generazioni. Noi non leggiamo nessuna valorizzazione del percorso d'istruzione tecnica, questo è il punto. Signor Presidente, tramite lei lo dico anche al senatore Lombardo. Noi abbiamo creduto e crediamo fino in fondo nella riforma del percorso tecnico professionale. Abbiamo creduto negli ITS e continuiamo a credere nel fatto che vada valorizzato tutto questo percorso. Qui, non leggiamo questa capacità di valorizzazione. Per questo abbiamo contestato l'accelerazione impressa dal Ministro a tutta la discussione avviata e in corso su tale provvedimento, nel momento in cui il disegno di legge arrivava come collegato al bilancio, con un ritardo rispetto ai tempi annunciati, ad un esame parlamentare che avrebbe richiesto un confronto più ampio tra le forze politiche.

avremmo dovuto audire di più il mondo della scuola, magari anche quelle realtà che avevano già partecipato alle precedenti sperimentazioni. Il Governo ha imposto un'accelerazione, non necessaria e imprevista. Soprattutto, mentre noi stavamo discutendo in Commissione, è entrato a gamba tesa, nel dibattito tesa, nel dibattito parlamentare in corso, con una circolare, che ha anticipato in gran parte i contenuti della riforma, adottata in virtù di un decreto ministeriale che, tra l'altro, ha ricevuto, come qui è stato ricordato in vari interventi, un parere negativo con osservazioni motivate da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In particolare, la sperimentazione è stata definita, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, frettolosa, priva del tempo necessario per orientare gli studenti e per formare e affiancare i docenti, perché non c'è nessun serio monitoraggio delle sperimentazioni già avvenute. Voglio ribadire che noi non abbiamo fatto nessuna discussione ideologica sulla quadriennalità.

ma andrebbero capiti e analizzati nel merito, non solo dal punto di vista quantitativo. Invece, noi abbiamo assistito a forzature, anche sui consigli di quelle scuole che dovevano aderire entro gennaio per poter avviare queste sperimentazioni Quindi, si è proceduto ad aggiungere un'altra sperimentazione, che comprime in quattro anni quello che è un percorso di cinque, senza intervenire in alcun modo sui *curricula*, sulle modalità di insegnamento e su come questo debba avvenire. Non vi sono fondi e questo aspetto risulta fondamentale per una riforma così ambiziosa, in cui si anticipano le esperienze lavorative

Ma che qualità di manodopera pensiamo di formare così? Quale dote formativa intendiamo dare alle ragazze e ai ragazzi? Io questo lo chiedo anche al mondo dell'impresa, che è così interessato a questo percorso. Che cosa chiedete? Che cosa si deve fare, se si vuole davvero riformare e rilanciare il settore dell'istruzione tecnica? Impostare una didattica per competenze, capace di affrontare la sfida di un nuovo percorso di studi, cambiando metodologia, affiancando i docenti e formandoli per quella che è una sfida educativa importante. Il lavoro è un contenuto educativo e noi questo lo riconosciamo. Ve lo dice una persona che ha amato un grande romanzo di Primo Levi, «La chiave a stella». Non c'è nessun disprezzo per il percorso tecnico. Anzi, c'è la preoccupazione che noi non diamo abbastanza forza a questo percorso e non favoriamo un adeguato orientamento degli studenti per avvicinarli ad esso. Non ci sono fondi. Gli stessi fondi previsti a sostegno dei *campus*, a seguito del passaggio in Commissione, sono dedicati a interventi infrastrutturali, non ad azioni dirette alle finalità sopra individuate. Siamo dentro un quadro confuso e l'abbiamo detto in più modi. Non abbiamo individuato in modo chiaro gli obiettivi curriculari e formativi da realizzare ed attuare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Questo vi chiedevamo e oggi l'abbiamo richiesto con i nostri emendamenti e con i ripetuti interventi della senatrice Malpezzi, sostenendo anche quelle parti del Paese *(Applausi)* in cui la realtà dell'istruzione e della formazione professionale è più indietro e il sistema degli ITS è meno diffuso e competitivo. Questa è la sfida e questa riforma non è all'altezza della sfida; rischia di perpetuare le differenze e i divari che già ci sono, di abbassare la qualità dell'istruzione tecnica e professionale, di disperdere le buone prassi e le competenze. Questo è l'altro punto essenziale per noi: le diseguaglianze che questo disegno di legge accentuerà. Si crea un canale separato per un'istruzione di secondo livello, tutta finalizzata a professionalizzare e piegare alle esigenze del mondo dell'impresa territoriale qui ed ora, senza fornire competenze adeguate e con differenze territoriali che aumenteranno le diseguaglianze di opportunità, segnando nelle differenze territoriali non capacità di promozione di risorse e sviluppo dei luoghi, ma destini diversi. *(Applausi)*. Del resto, l'avete già scelto con l'autonomia differenziata. Per noi non è questo il ruolo dell'istruzione tecnica e professionale nel nostro Paese e riteniamo in linea con gli obiettivi posti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che la stessa vada valorizzata e potenziata con pari dignità rispetto ai percorsi di istruzione liceale; valorizzata e promossa con risorse e strumenti adeguati, in un'ottica sempre formativa e non meramente professionalizzante, nel contesto di un quadro produttivo in costante e continua trasformazione, che richiede un di più di competenze, un di più di istruzione in una prospettiva nazionale e non solo centrata sulle peculiarità, le caratteristiche e le esigenze dei singoli territori coinvolti. Sarebbe invece necessario - l'abbiamo ribadito - individuare delle linee guida altrimenti corriamo il rischio (e questa contrarietà a linee guida generali è frutto di questo) di una destrutturazione. Non è un giudizio ideologico, ma è un giudizio che fa fede della discussione che abbiamo avuto in Commissione e oggi in Aula: di una destrutturazione del sistema nazionale di istruzione, anche rispetto alla predisposizione dei curricoli, che viene di fatto consegnato al governo delle reti, che diventeranno il soggetto di riferimento delle Regioni. Troviamo questa impostazione sbagliata. Bisognerebbe costruire, a partire dal rilancio dell'autonomia scolastica, che ne è punto di forza indispensabile, un progetto educativo e territoriale che comprenda e sviluppi anche l'educazione permanente degli adulti, ma vedere nel territorio solo un mercato economico a chilometro zero significa mortificarne il potenziale educativo *(Applausi)* e nello stesso tempo privare le istituzioni scolastiche di una risorsa fondamentale per rendere il proprio piano dell'offerta formativa lo strumento capace di indurre negli studenti e nelle studentesse quella riflessione sulla realtà in cui vivono e di cui hanno profondo bisogno. Noi non vediamo sinergia; anzi, avremmo voluto una sinergia col mondo produttivo. Noi vediamo il rischio di una scuola piegata alle esigenze contingenti del mondo produttivo non ci sorprende in un Governo che non ha politiche industriali, che sta svendendo *asset* significativi di questo Paese. *(Applausi)*. Non c'è l'idea che la formazione tecnica e professionale sia una leva di cambiamento e di sviluppo diverso, investendo sulla forza lavoro e sulle necessità formative dei ragazzi e le ragazze. È per questo che voteremo contro questa riforma, calata dall'alto sul mondo della scuola. Per questi motivi dichiaro il voto contrario del Gruppo Partito Democratico.

desidero, in premessa di questo mio intervento, innanzitutto ringraziare la relatrice, la collega senatrice Bucalo, per le consuete capacità e puntualità nel lavoro svolto prima in Commissione, poi in Aula, così come desidero ringraziare il presidente della 7a Commissione permanente, senatore Marti, e tutti i colleghi della Commissione per il grande clima di confronto, sempre diretto ma garbato, che anima le nostre discussioni e la conduzione dei lavori. Naturalmente, saluto e ringrazio il Governo, qui rappresentato dalla autorevole presenza del sottosegretario Frassinetti. Quello di oggi è un ulteriore tassello nella costruzione di una politica figlia di una visione nuova che vogliamo portare e realizzare facendo in modo che la formazione scolastica sia in dialogo con la formazione professionale e con il mondo delle imprese, che evidentemente è quello che per troppo tempo è mancato, se nell'ultima indagine di Unioncamere e ANPAL risulta che su 508.000 assunzioni programmate dalle imprese ben 250.000 sono rimaste inevase per mancanza di candidati oppure per la presenza di candidati con una preparazione insufficiente. Basterebbe solo ed esclusivamente questo per dire che evidentemente chi ha mosso delle critiche dovrebbe almeno farsi animare da qualche dubbio rispetto alla propria visione che è stata in campo fino a circa quattordici mesi fa e che consegna una fotografia che è esattamente nei numeri che ho letto.

ho ascoltato dichiarazioni che hanno un sapore esclusivamente ideologico e che appartengono a quella visione che o poteva fare e non ha fatto, o che evidentemente dovreste mettere in discussione se questi sono i dati. Peraltro, con questo provvedimento realizziamo l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in tal modo contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione. Come ha detto probabilmente in parole più semplici delle mie il presidente Marti, qui non si toglie nulla a nessuno, anzi si aggiunge una possibilità. Parlare di frammentazione guardando l'attuale e complessivo sistema significa che evidentemente siete affezionati all'inerzia. Dire che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi significa iscriversi ad una visione antiquata che non parte dalla constatazione di realtà, di quello che è il mondo della formazione. Vorrei rivolgermi alla senatrice Malpezzi, verso la quale

per fare in modo che questa propensione trovi rispondenza in un suo compagno di partito e di corrente, il governatore della mia Regione,

e di fare in modo che non si pensi a fare battaglie politiche per l'affermazione della propria personalità e della propria carriera sulle spalle di giovani, di studenti e di territori che hanno tanto da dire in termini di *made in Italy* e che hanno tanto da rappresentare in termini di racconto dell'italianità.

la seconda realtà in Europa in termini manifatturieri. Noi vogliamo che il nostro futuro sia scritto agganciandoci alla tradizione delle nostre radici; vogliamo fare in modo che ci sia possibilità e capacità di scegliere, di avere reali opportunità per un futuro; tuttavia dobbiamo anche dirci, in assoluta onestà, che in quel sistema della formazione professionale che veniva richiamato

potevano trovare un lavoro, ma non lo hanno trovato. Noi, invece, attraverso questi provvedimenti, vogliamo produrre occupati reali, persone che ricavano la dignità e l'onore delle proprie esistenze dal lavoro. *(Applausi)*. Ho sentito anche questioni che non c'entrano assolutamente nulla con il provvedimento in discussione. sentito parlare dei certificati di collaudo sulla staticità degli istituti. Se vogliamo andare fuori tema, facciamolo, me lo concedo anch'io e vi invito a vi invito a leggere i rapporti dell'Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola che, dal 2018 al 2021, cioè quando avete governato voi,

gli stessi istituti si trovavano nella stessa percentuale (50 per cento), quindi non avete fatto assolutamente nulla

che tirano in ballo l'etnia, come se gli italiani dovessero svolgere soltanto professioni di carattere intellettuale, mentre poi per la manovalanza ci sono gli immigrati che noi non vogliamo in Italia. *(Applausi)*. La vostra è una visione profondamente discriminatoria. Noi diciamo che il lavoro, qualunque tipo di lavoro fatto in maniera onesta, competente e con dedizione, sosteniamo che tutti devono avere la possibilità di poter esprimere la propria personalità e le proprie inclinazioni, ma dobbiamo leggere anche la realtà. Pensare ancora a un mondo in cui c'è separazione tra il mondo della scuola, il mondo della formazione professionale e le imprese è qualcosa che appartiene letteralmente al secolo scorso. una contrapposizione e un lavoro per compartimenti stagni che ha determinato il fallimento che noi oggi abbiamo raccolto e che, con il voto degli italiani, vogliamo assolutamente cambiare.

per il 2025 e il 2026. Colleghi, credo che questa sia un'occasione persa per chi non esprime un voto favorevole su questo provvedimento. Noi lo faremo in maniera convinta perché, se la realtà grida, voi avete deciso di fare un processo alle intenzioni, mentre noi abbiamo deciso di non lasciarla gridare nel vuoto.

sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026"; sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".

vota. Non funziona così. Sembra un emendamento più che un coordinamento formale. Se cambiano gli anni, c'è scritto un anno e diventa un altro anno, è un'altra legge e non un coordinamento formale. modifiche arrivano in diretta. Vorrei chiederle, Presidente, di passare la seguente informazione al presidente La Russa: almeno una parte di questo Senato ambirebbe a leggere le cose che vota in precedenza. È infatti il secondo accadimento della giornata. Mi perdoni, leggo in diretta con lei. Sostituire le parole «2023-2025» con le seguenti «2024-2026» le sembra un coordinamento formale? A me sembra che stia cambiando l'ambito di applicazione temporale della legge. Sono incredulo. Abbiamo assistito a pause perché la maggioranza non aveva l'accordo. Abbiamo assistito al cambiamento di pareri in corsa e ora cambiamo anche l'ambito di applicazione temporale della legge. Sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per l'anno 2024": c'è anche proprio un tema di contabilità - non lo so - di ambito

Io credo che siamo fuori tempo massimo, perché abbiamo votato gli emendamenti, abbiamo sentito le dichiarazioni di voto finali e dobbiamo votare il disegno di legge

testo che è stato distribuito adesso viene considerato coordinamento formale del testo e, all'articolo 2, dice di apportare modifiche. Quest'altro invece è l'emendamento 4.1000, presentato dalla relatrice, identico al coordinamento formale del testo. Quindi qui era un emendamento, che è stato votato e approvato alcuni minuti fa come emendamento all'articolo 4. Ora invece viene presentato come un coordinamento formale del testo. Allora, ci spiegate se è un emendamento? *(Applausi)*. Insomma, una volta è emendamento e una volta è coordinamento del testo.

all'articolo 4. Non si capisce perché la relatrice non sia stata in grado di farlo nella fase precedente anche per quanto riguarda l'articolo 2, se non altro per portare le modifiche. Ma il tema è che questo è un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento. Lo so che questa non è la giornata giusta per fare domande, perché nessuno ci vuole rispondere. Ma il tema di fondo è il la legge di bilancio aveva votato all'interno del provvedimento in un determinato modo, questo modifica la legge di bilancio e di conseguenza altro che coordinamento formale dei testi. *(Applausi)*.

di norma, appunto, il coordinamento formale si ha su piccoli aspetti e non su temi che cambiano gli aspetti temporali di un provvedimento. Signora Presidente, qui veramente sembra che, ricostruendo i pezzi, la situazione si aggravi vieppiù. Prima scopriamo che un emendamento identico è un emendamento - come ha appunto ricordato il senatore De Cristofaro - e quindi viene votato in quanto tale; poi invece lo stesso emendamento viene presentato come coordinamento, per cui non c'è bisogno di ricominciare la procedura e di far esaminare all'Assemblea il provvedimento, così come necessario. La soluzione sarebbe piuttosto semplice, se ci fosse il rispetto delle istituzioni. Si manda il provvedimento alla Camera, lo si modifica in seconda lettura e torna al Senato. È molto semplice!

ingolfiamo gli uffici di decreti su decreti, a botta di due o tre decreti alla settimana, questo poi provoca delle sviste e può provocare degli errori. Quindi, davvero chiediamo al Governo di avere più rispetto per il Parlamento, di rallentare, di prendere un attimo di respiro,

apportare le seguenti modificazioni:* sopprimere le parole: "delle proiezioni"; sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026"; sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024". *Allegato

Il Senato non è in numero legale.

i cori mi sembrano eccessivi in ogni occasione.

intervengo solo per consigliare, attraverso di lei, ai colleghi Presidenti dei Gruppi di maggioranza di chiuderla qui per oggi, perché è uno spettacolo penoso che quest'Aula non merita. *(Applausi)*. È evidente che un provvedimento vuoto - era vuoto, come abbiamo detto più volte in tutti gli interventi - viene definitivamente

Io invece, prima di apprezzare le circostanze, ritengo che sia importante che il Senato dimostri se è in grado di avere il numero legale e, quindi, sospendo la seduta

*(IV-C-RE)*. Signor Presidente, esattamente trent'anni fa il Parlamento della Repubblica varava la legge nazionale della montagna, una iniziativa legislativa importante che arrivava alla fine di un percorso storico, peraltro significativo. Fu una delle ultime leggi della cosiddetta Prima Repubblica. Gli alfieri del cambiamento e della trasformazione che arrivarono dopo non produssero nulla che potesse sostituire questo strumento che, per alcuni aspetti, ha ancora molti elementi di importanza. L'intera parte sui principi, ad esempio, è scritta in maniera assolutamente fondamentale. Per altri aspetti, la parte applicativa inseriva un meccanismo di sussidiarietà che consentiva la valorizzazione dei Comuni e delle comunità montane nel quadro di una legislazione regionale ancora incipiente e, sul piano dei contenuti più specifici, introduceva una serie di misure che voleva rendere concreto uno *slogan* all'epoca abbastanza frequente e, cioè, la montagna risorsa e non problema. Dopo trenta anni e dopo tanti tentativi di riforma, tutti regolarmente non arrivati in fondo, crediamo che si debba - da un lato - sottolineare l'importanza di questo momento e - dall'altro lato - recuperare quello spirito per assicurare ad una parte significativa del nostro territorio nazionale, peraltro tutelata e sancita dall'articolo 44 della Costituzione, di avere finalmente una legge nazionale che sia all'altezza dei tempi che sono cambiati. Il modo migliore per ricordare questo trentennale, oltre che ringraziare le donne e gli uomini che lavorarono a questo significativo risultato, è aprire una stagione riformatrice che vada nella direzione di assicurare pari dignità e tutela a un territorio che si sta spopolando sempre di più, che sta vedendo un invecchiamento della popolazione

personalmente nei primi anni della mia attività professionale di avvocato. Ne ho un ricordo stupendo, anche per la sua giovialità, il suo carattere e il suo modo gioioso di affrontare la vita. *(Applausi)*. Prego, «sarà per quella faccia mite, da primo della classe che si lascia copiare i compiti, sarà per il rigore che dimostra nelle sue inchieste, Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare perché non combina sciocchezze». Signor Presidente, senatrici, senatori, scriveva così sulle colonne del «Corriere della Sera» Walter Tobagi il 29 gennaio 1979 all'indomani dell'agguato compiuto a Milano da un gruppo di fuoco di Prima linea a danno del giudice Emilio Alessandrini. Due giorni fa, il 29 gennaio, abbiamo ricordato questo servitore dello Stato a quarantacinque anni da quell'attentato che gli rubò la vita; una vita dedicata alla ricerca della verità e della giustizia, con un impegno senza riserve su alcune tra le inchieste giudiziarie più complesse e delicate della storia della Repubblica. Con la sua competenza, la sua integrità e la sua passione seppe affrontare le sfide più difficili senza mai cedere alle pressioni, alle intimidazioni e alle minacce. Furono questi motivi per cui Alessandrini divenne un bersaglio per chi voleva colpire il cuore della democrazia; un bersaglio da colpire proprio mentre si recava al lavoro, quel giorno, così tanto amato e onorato del suo impegno. «Uno dei magistrati che maggiormente ha contribuito in questi anni a rendere efficiente la procura della Repubblica di Milano»; queste le parole utilizzate nel documento di rivendicazione di Prima linea, eloquenti delle presunte colpe che la follia terroristica addebitava al giudice. Nato e cresciuto in Abruzzo, Emilio Alessandrini, dopo gli studi a Napoli, aveva avviato la sua carriera in magistratura con il primo incarico presso la procura di Bologna nel 1967. Già nel 1968 passerà a nuovo incarico presso la procura della Repubblica di Milano nel ruolo di sostituto, ufficio per il quale si guadagnerà grande stima e reputazione. Basti pensare che già nel 1971 il consiglio giudiziale di Milano, nell'esprimere parere favorevole alla nomina di aggiunto giudiziario, sottolineerà come in soli il sostituto procuratore sia stato in grado di definire 687 procedimenti, partecipato a 116 udienze e redatto 97 requisitorie, ritenendo doveroso porre in rilievo lo zelo encomiabile, la marcata marcata capacità dialettica, la profondità di indagine e il perfetto equilibrio del dottor Alessandrini. Questa prima fase del suo lavoro è caratterizzata da inchieste sull'eversione di destra, particolarmente preoccupante nell'Italia di quegli anni a Milano, per mano delle SAM (Squadre d'azione Mussolini), responsabili di atti dimostrativi e dinamitardi. Il giudice non sarà affrancato dalle azioni del gruppo terroristico. Un ordigno infatti sarà fatto esplodere nell'immobile in cui risiedeva con la sua famiglia, senza fortunatamente causare vittime, ma a fine intimidatorio. Sono anche gli anni dell'inchiesta su Piazza Fontana, che il giudice seguirà con attenzione e scrupolo. Ed è proprio su questa istruttoria che il lavoro di Alessandrini si incontrerà con quello di altri compianti e autorevoli magistrati: anzitutto il giudice Occorsio, anch'egli vittima del terrorismo nero nel 1976, che per primo si occupa del caso, ottenendo a Roma il rinvio a giudizio della anarchico Valpreda e del neofascista Stefano Delle Chiaie. la seconda istruttoria sulla cosiddetta pista nera, ottenendo il rinvio a giudizio della cellula fascista veneta nel 1974, lavoro successivamente portato a termine da un altro giovane magistrato, Gherardo D'Ambrosio. Saranno anni di grande impegno anche sull'eversione di estrema sinistra, in particolare sull'autonomia operaia milanese, nonché sulle vicende riguardanti il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, indagine che non riuscirà a proseguire a causa del piombo terroristico. anni da quel tragico evento, vogliamo rendere omaggio a questo eroe civile, che ha sacrificato la sua vita per i valori in cui credeva. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il suo lavoro, che ha contribuito a svelare la verità su fatti oscuri e a far luce su trame criminali... sua eredità, che è quella di una magistratura indipendente, efficiente, al servizio di cittadini e della Costituzione. Emilio Alessandrini è un esempio per tutti noi, che ci ispira a non rinunciare mai alla nostra dignità e ci ricorda che il prezzo della libertà è l'impegno civile, così come il dovere della democrazia. Fu il primo magistrato ucciso dal terrorismo rosso a Milano e la sua morte sconvolse la città e il Paese intero. I funerali saranno un tributo di popolo, con più di 200.000 persone in Piazza Duomo. "La solidarietà del popolo alla magistratura dimostra che il terrorismo è un fatto isolato": con queste parole l'indimenticato presidente della Repubblica Pertini renderà omaggio al trentaseienne giudice assassinato. Con lo stesso doveroso impegno istituzionale, Presidente, e con lo stesso spirito di riconoscenza oggi in quest'Aula rendiamo onore alla sua memoria. Un abbraccio da qui alla sua famiglia, alla moglie Paola, al figlio Marco; gratitudine e riconoscenza a chi in questi giorni ha doverosamente promosso il ricordo del giudice. Grazie al Comune di Milano e al sindaco Sala. Grazie al Comune di Pescara e al Consiglio superiore della magistratura...

i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera. È stato un lavoro che la Commissione affari esteri ha portato avanti per diverso tempo e che ha visto anche scontrarci sul telelavoro e su altre a seguito di questo accordo è stato rivisto l'elenco dei Comuni che ricadono nei 20 chilometri per essere considerati frontalieri tra Italia e Svizzera.

tra Italia e Svizzera, il nuovo elenco di Comuni che ricadono nei 20 chilometri ha portato però a considerare i frontalieri già esistenti, ricadenti nei nuovi Comuni considerati, a vedersi scrivere dalla Dipartimento delle finanze e dell'economia della divisione delle contribuzioni del Canton Ticino che in realtà per loro non vale l'accordo, in quanto considerati nuovi frontalieri. Si parla dei Comuni di Misinto, Cogliate, Lentate, Barlassina e Meda. È un elenco piuttosto nutrito e lungo, che porterà questi lavoratori, che già erano frontalieri, a vedersi considerati nuovi frontalieri e avere la doppia imposizione, che invece l'accordo prevedeva fosse tolta. Io chiedo quindi al MEF che si attivi per verificare con le autorità svizzere affinché i vecchi frontalieri vengano considerati frontalieri alla stregua degli altri che già lo erano.